In merito alla questione delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, rammento che l'accesso alle cure previste nell'ambito dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) è sempre garantito agli assistiti agli assistiti iscritti al Servizio sanitario nazionale, sia pure non in esenzione, secondo criteri di efficacia e di appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali. In particolare, le prestazioni di riabilitazione sono incluse nei LEA e la loro erogazione demandata alla competenza delle singole Regioni attraverso le Aziende sanitarie locali. L'emergenza di impedimenti nell'erogazione può essere ascritta a difficoltà organizzative regionali e locali. Nel merito della questione posta, si osserva che la dispensazione delle guaine elasto-compressive è prevista dall'allegato 5 del 12 gennaio 2017, recante la definizione e l'aggiornamento dei LEA, la cui effettiva entrata in vigore, tuttavia, resta condizionata alle disposizioni finali e transitorie dello stesso che prevedono l'adozione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di definizione delle tariffe delle medesime prestazioni. Va anche detto che le disposizioni che regolamentano l'accesso degli assistiti al Servizio sanitario nazionale non prevedono il rimborso a posteriori di prestazioni erogate in ambiti privati, tanto più se non incluse nei LEA. La stessa direttiva n. 24 del 2011del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, prevede il rimborso di prestazioni erogate all'estero, nell'Unione europea, anche da strutture private, purché ricomprese nei LEA. Concludo rassicurando la senatrice interrogante che sarà impegno del Ministero della salute, attesa la rilevanza della questione in esame e in considerazione delle legittime aspettative dei pazienti coinvolti, compatibilmente con le attività finalizzate a fronteggiare l'emergenza in corso, garantire in tempi rapidi, mediante la definizione delle tariffe di cui sopra, la dispensazione delle guaine elasto-compressive.

aggiungo due elementi. Il primo è che sarà mia premura favorire lo sviluppo di una rete territoriale, che manca fondamentalmente, soprattutto quando si parla di malattie rare. I pazienti e le famiglie spendono soldi per muoversi e hanno problemi con il lavoro, perché spesso non sanno dove andare. andare. È sicuramente necessaria una migliore circolazione delle informazioni e chi meglio del Ministero, nel suo sito e nella sua sede, può aiutare a farle convogliare e ridistribuirle in periferia? Allo stesso modo, in periferia è necessario che vengano resi univoci i percorsi clinici e diagnostici di presa in carico, cura e riabilitazione, affinché in tutto il Sistema sanitario nazionale - e, quindi, nelle varie Regioni - vi sia un'uniformità di cure. cure. Sarà mio impegno far sì che questa rete porti fiducia, protezione e sicurezza per gli operatori (che si occupano di linfedemi primari, entrino in comunicazione con coloro che soffrono di linfedemi secondari, e quindi ci possa essere uno *share* di informazioni che si traduca in sicurezza per gli operatori e, ancor di più, per i

signor Vice Ministro, visto che ne abbiamo parlato molte volte, che siamo in attesa di due importanti punti di riferimento. Da un lato, la pregherei di accelerare, presso la Camera dei deputati, l'approvazione del disegno di legge sulle malattie rare.

Dobbiamo aumentare il livello di conoscenza delle malattie rare attraverso sia il *curriculum* di studi ordinari della Facoltà di medicina, sia le diverse branche specialistiche. Questo è il primo punto. L'ignoranza che il medico ha nei confronti della patologia aggiunge frustrazione a frustrazione per il malato.

veramente cari: nel momento in cui il paziente non può permetterseli, diventano discriminanti rispetto alla qualità della salute (cosa che non vogliamo, proprio perché il nostro sistema sanitario nazionale è gratuito e universalistico). Perché i pazienti devono o cercano di accedere al privato per avere la prescrizione? Semplicemente perché nel pubblico non trovano, in quel momento, la conoscenza del problema, la sensibilità verso la malattia e la tempestività nella risposta.

che siano l'analogo di un farmaco salvavita, però lo diventano di un farmaco fondamentale per la qualità della vita di questi pazienti. Dobbiamo assolutamente riuscire a facilitare il paziente, affinché non abbia problemi nel momento in cui ha bisogno della guaina, esattamente come un paziente portatore di una qualsiasi disabilità non deve avere problemi,

per cui auspichiamo che il Ministero riassuma tale competenza). Ora, nel caso delle malattie rare, abbiamo bisogno di una cabina di regia forte nel Ministero e poi di centri specialistici a livello regionale. Questo sistema, che chiamiamo *top-down*, rientra nella sua responsabilità. Quindi tra sei mesi ripresenterò la stessa interrogazione e, nel frattempo, gliene presenterò puntualmente altrettante per tante malattie rare e per tanti malati rari che aspettano una risposta. *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*.

Presidente, onorevoli senatori, la problematica evidenziata dagli interroganti è da tempo all'attenzione del Governo e di questo Ministero, stante l'obiettivo di predisporre un pacchetto di misure volte a rendere più incisivi gli strumenti di contrasto all'incremento delle popolazioni di ungulati selvatici, a cui deve ora essere data concretezza anche attraverso una modifica della legge n. 157 del 1992. Evidenzio tuttavia che, a fronte delle competenze regionali in materia, alcune Regioni stanno regolamentando il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157 del 1992, attraverso la predisposizione,

Sempre a tal proposito, ricordo che è all'esame della Camera dei deputati la proposta di legge n. 982, recante disposizioni di sostegno e di semplificazione per il comparto agricolo, che introduce misure volte ad agevolare ulteriori interventi di contenimento, tra cui l'ampliamento dell'arco temporale nel quale è autorizzata la selezione. In accordo con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato istituito un gruppo di lavoro incaricato di formulare proposte per l'adeguamento del quadro normativo e sanzionatorio relativo ai danni da fauna selvatica, che ha presentato una relazione conclusiva contenente talune linee di intervento attualmente all'attenzione dei Ministri competenti. Tra le proposte avanzate, tenendo anche conto dell'esigua consistenza di personale delle amministrazioni regionali e provinciali, si è evidenziata la necessità che anche altre figure specializzate vengano autorizzate a effettuare attività di controllo numerico delle specie faunistiche, attraverso coadiutori formati mediante appositi corsi validati dall'ISPRA. Quanto sopra appare altresì funzionale alla finalità di dare effettiva applicazione al Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia e Piano di eradicazione in Regione Sardegna per il 2020, predisposto dal Ministero della salute e volto a proteggere il patrimonio suinicolo nazionale dal rischio di trasmissione del virus della peste suina. Per quanto riguarda poi le problematiche relative al risarcimento dei danni del settore agricolo, quest'amministrazione ha provveduto a effettuare la notifica alla Commissione europea di uno schema di decreto interministeriale che disciplina le modalità di concessione degli aiuti per le misure preventive e per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, secondo le indicazioni e i criteri indicati dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e delle zone rurali per il periodo 2014-2020. Con decisione C(2019)8522 finale della Commissione europea del 21 novembre 2019 è stato approvato tale regime di aiuti. Il citato decreto prevede infatti la possibilità di risarcimento dei danni alle sole imprese attive nella produzione agricola primaria, arrecati ad attrezzature e infrastrutture animali da qualsiasi animale che risulti protetto dalla legislazione unionale o da quella nazionale, considerando così anche specie diverse da quelle individuate dalle direttive Habitat e Uccelli esempio il cinghiale e altre specie cacciabili), i cui danni possono essere compensati, purché si verifichino sul territorio di un'area protetta. Per quanto concerne invece i danni provocati da animali non protetti in aree in aree esse stesse non protette, è possibile soltanto un indennizzo attraverso gli aiuti in regime *de minimis*. In tale ambito, a seguito della modifica del regolamento UE 1408/2013, il limite agli aiuti in regime *de minimis* per impresa è stato innalzato a 25.000 euro.

per far fronte ai danni causati dalla fauna selvatica si ritiene dovrà essere valutata in relazione alle diverse priorità d'intervento e alla sua compatibilità con le esigenze di finanza pubblica.

di pervenire alla definizione di un nuovo quadro normativo in materia, in grado di tutelare l'incolumità pubblica e le produzioni agricole.

la solidarietà e la vicinanza di noi presenti al senatore e nostro segretario federale Matteo Salvini per quanto accaduto ieri a Pontassieve in Toscana, dov'è stato aggredito nel corso di un'attività democratica d'incontro con i cittadini. Mi permetta di dire basta a questi odiatori seriali, che combattono i nemici politici non con le idee e con le proposte, ma con la violenza, che va sempre condannata, soprattutto da quest'Assemblea. Il miglior commento l'ha fatto lo stesso Matteo Salvini pochi minuti dopo: alla rabbia di pochi rispondiamo con il sorriso, il lavoro e la speranza di tanti. Lo condividiamo e applaudiamo anche a questa riflessione

i lupi di oltre il 650; l'incremento delle predazioni da parte di questi ultimi, dei carnivori, sta mettendo a dura prova l'allevamento di carattere familiare. È notizia di questi giorni il dramma che sta vivendo una provincia come quella di Belluno, dove addirittura una delegazione guidata dal mio collega Paolo Saviane è stata dal prefetto per illustrare la pericolosità per la vivibilità e per il lavoro su quel territorio. Bisogna intervenire subito; se non volete ascoltare noi che siamo l'opposizione, ascoltate le istituzioni locali, perché sono fondamentali. Per quanto riguarda nello specifico i cinghiali,

Oltre 20 persone sono decedute in seguito a questi incidenti. Oggi si stima la presenza in Italia di oltre due milioni di esemplari di cinghiali, con 200 milioni di euro annui di danni complessivi.

però non c'è nulla di operativo: i risarcimenti devono essere fatti. Le Regioni si stanno attivando singolarmente, ma questo non va bene; ci dev'essere una regia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

anche a livello selettivo, come ha detto, ma la regia dev'essere nazionale, perché, se si lascia la potestà a ogni singola Regione, ce ne sono alcune che non intervengono affatto e questo è drammatico, come sa meglio di me.

Dica al ministro Bellanova che prima dei clandestini vengono gli agricoltori italiani, che soprattutto vogliono risposte immediate e certe.

che all'interno della pubblica amministrazione, agli alti livelli nazionali e regionali - ho avuto confronti sul tema - ci sono persone che conoscono la realtà, che non è quella pensata da coloro che vivono nei salotti e non hanno mai visto un cinghiale o un lupo dal vivo.

La Provincia di Cuneo ha 17 guardie venatorie e della pesca che, una volta esperite le funzioni d'ufficio, tenuto

Signor Presidente, onorevoli senatori, con riferimento ai fatti esposti, si rappresenta che il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza pubblicata il 23 dicembre 2019, n. 8693, ha respinto il ricorso in appello delle amministrazioni governative regionale per il Lazio n. 72 del 2019 e ha accolto l'appello incidentale dell'architetto Giuseppe Leoni, sancendo il principio per cui «alle amministrazioni governative titolari di tale potere non residua alcuna discrezionalità, una volta constatato che l'originario ricorrente è in possesso dei requisiti previsti per la nomina e che il procedimento di designazione di competenza dell'assemblea dell'Aereo Club d'Italia si è svolto legittimamente». La suddetta sentenza ha inoltre ordinato alle amministrazioni ministeriali appellanti di nominare l'architetto Giuseppe Leoni presidente dell'Aero Club d'Italia, laddove non ricorrano le circostanze ostative, con riferimento al possesso dei requisiti soggettivi previsti, sia di ogni altro eventuale profilo di legittimità, intimando a formulare formulare proposta, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53. La Corte d'appello di Roma, terza sezione penale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto l'architetto Giuseppe Leoni dal reato ascritto, annullando la sentenza del tribunale penale di Roma del 14 dicembre 2016, perché il «fatto non costituisce reato», con dispositivo di sentenza reso pubblico in udienza in data 11 giugno 2019. A carico dell'architetto Giuseppe Leoni erano stati iscritti altri tre procedimenti penali, in parte aventi ad oggetto gli stessi fatti di cui sopra, tutti definiti con decreto di archiviazione a seguito di relativa richiesta. Si segnala, inoltre, che la Corte dei conti ha assolto l'architetto Giuseppe Leoni con sentenza n. 355 dell'11 luglio 2019, mentre nulla risulta in ordine ad ulteriori irregolarità che sarebbero state accertate dal Commissario straordinario dell'ente. Pertanto, in ottemperanza della sopra accennata sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 8693 del 2019, non essendo state ravvisate motivazioni ostative, è stato dato seguito, per il periodo residuo, alla delibera assembleare dell'ente n. 5 del 2017, con cui l'architetto Giuseppe Leoni è stato designato ai fini della successiva nomina di presidente dell'Aero Club d'Italia, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53. In data 17 giugno 2020 è stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina dell'architetto Giuseppe Leoni quale presidente dell'Aero Club d'Italia, registrato dalla Corte dei conti in data 15 luglio 2020, con foglio n. 1602.

Su questo pesa, *in primis*, il giudizio relativo al ritardo che registra tale risposta ad un atto presentato un anno fa. Nelle more, come lei ha detto, signor Sottosegretario, è stato nominato di nuovo il presidente dell'Aero Club d'Italia nella persona dell'architetto Leoni, che è parte centrale della questione. Quindi la mia perplessità, rispetto alla soddisfazione assolutamente parziale, insiste sul fatto che permane evidente una contraddizione che lei oggi - mi dispiace dirlo - non ha saputo risolvere. Le motivazioni gravi, serie e importanti contenute nel decreto del faccio riferimento ad esempio a quello di nomina del commissario Valori - ed espresse dai Ministeri vigilanti per i quali si ravvisano problemi legati alla eleggibilità dell'architetto Leoni, sono ancora valide e tutte sul tappeto. Alcuni tra i fatti contestati, come la concessione di incarico di elevata professionalità in contrasto con il contratto collettivo nazionale di lavoro, o ancora la nomina a direttore generale a vantaggio di persona con età superiore ai limiti previsti per il collocamento dei pubblici dipendenti anni), o ancora una serie di atti che, stando alle date di nomina, risultano nulli perché deliberati da organi ormai decaduti, certamente non possono non incidere nella scelta di chi è chiamato a presiedere un ente di diritto pubblico. Per questo - lo ribadisco - sono assolutamente insoddisfatto della risposta, ma mi aspetto anche una presa di posizione del Ministro, perché credo che su un organo come quello per il quale l'architetto Leoni è chiamato ad una funzione importante il Ministro possa e debba dire qualcosa di più.

Presidente, onorevoli senatori, le misure adottate dal Governo volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno avuto, e in parte continuano ad avere, ripercussioni in particolare sugli adolescenti e sui bambini, privati improvvisamente della possibilità di andare a scuola, di avere relazioni sociali e di fare sport. Con riferimento al primo quesito, è allo studio una proposta normativa volta a promuovere il coordinamento delle politiche giovanili fra i diversi livelli di governo, nel contesto delle politiche e delle azioni previste dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa, assicurando la partecipazione attiva dei giovani compresi tra i quattordici e i trentacinque anni di età nei processi decisionali e nelle scelte politiche che li riguardano, nonché di provvedere alla revisione organica della normativa in materia di servizio civile e del riordino della stessa al fine di razionalizzare le fonti e semplificare le procedure del servizio civile universale. Inoltre, è prevista l'istituzione di un tavolo nazionale per le politiche giovanili con funzione di indirizzo e concertazione nonché di monitoraggio e valutazione degli interventi nazionali e territoriali in favore delle giovani generazioni, funzionale alle attività di programmazione e pianificazione segnalate dall'onorevole interrogante. Il suddetto tavolo nazionale potrà fornire una risposta adeguata in termini di crescita e di realizzazione delle politiche orientate alle giovani generazioni che possano consentire di riaffermare la centralità dei giovani nelle scelte di crescita del Paese, attivando un sistema decisionale idoneo a cogliere le opportunità di sviluppo delle politiche giovanili mediante un raccordo ed un adeguamento costante anche con le iniziative sostenute nell'ambito dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa. Il tavolo, infatti, dovrebbe tra l'altro promuovere e favorire i processi di inclusione, autonomia, protagonismo e partecipazione attiva dei giovani al processo democratico di scelta politica e nella società civile. rappresenterebbe lo strumento di coordinamento dei vari *stakeholder*, utile a costruire interventi trasversali, organici e coerenti in materia di politiche giovanili, in termini sia istituzionali, sia tematici, sia geografici, evitando in tal modo sovrapposizioni, duplicazioni e diseconomie, in un'ottica di efficientamento della spesa e dei benefici ad essa sottesi. Tenuto conto che le decisioni adottate in termini di pianificazione e monitoraggio potrebbero incidere su interventi che rientrano nella sfera di attribuzioni delle Regioni e del sistema degli enti locali, oltre che dei vari Ministeri, si sottolinea la sua funzione di indirizzo, coordinamento e monitoraggio di una strategia sinergica e integrata in materia di politiche giovanili. Pertanto, l'obiettivo è che il tavolo costituisca uno strumento di condivisione in grado di promuovere diverse azioni, in accordo e collaborazione tra i vari soggetti titolari di politiche dirette e, in questa accezione, per la sua realizzazione realizzazione e attuazione dovrebbe fondarsi su un'attività di cooperazione istituzionale, che vede in primo piano il ruolo delle Regioni e del sistema degli enti locali. Relativamente al secondo quesito, si conferma che lo stanziamento per il 2020 del fondo per le politiche giovanili ha capienza per l'attivazione di una o più iniziative specificamente dedicate ai giovani, che potranno aggiungersi a quelle già avviate dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale negli anni passati in favore delle giovani generazioni e che risultano tutt'ora in corso attuazione. Si richiamano brevemente. In primo luogo, l'avviso pubblico «Prevenzione e contrasto al disagio giovanile», finalizzato al finanziamento di azioni volte ad intervenire su giovani in condizioni di disagio, favorendo l'inclusione e l'innovazione sociale. In particolare, si segnala l'ambito che riguarda la prevenzione e il contrasto al disagio giovanile attraverso la promozione di azioni di sistema sui territori che, mediante l'innovazione sociale dei lavori in rete, agiscono per contrastare l'esclusione e la diffusione di comportamenti a rischio, con riferimento all'individuazione e al reinserimento di giovani cosiddetti NEET l'avviso pubblico «Orientamento e *placement* giovani talenti» promuove azioni tese a sostenere l'inserimento lavorativo e l'autoimprenditorialità dei giovani talenti, attraverso iniziative innovative di orientamento e *placement*, a valere sulle risorse del fondo per le politiche giovanili. avvisi pubblici «Giovani per il sociale 2018» e «Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018»: si tratta di due avvisi pubblici finanziati nell'ambito del piano di azione e coesione (PAC) per il finanziamento di progetti presentati da giovani e organizzazioni del privato sociale e rivolti a giovani beneficiari in un'età compresa tra i quattordici e i trentacinque anni. I suddetti avvisi si inseriscono nel contesto delle azioni rivolte ai giovani del *non profit* per lo sviluppo nel Mezzogiorno. L'iniziativa, rivolta ai giovani *under* trentacinque del Sud Italia nell'ambito del piano di azione e coesione, è finalizzata a promuovere e a sostenere i progetti del privato sociale per il rafforzamento della coesione socioeconomica del Sud, mediante la creazione di reti in grado di leggere i bisogni emergenti e tradurli in proposte progettuali concrete, sostenibili ed efficaci. Vi è poi il bando «Fermenti», il bando «Fermenti», che rappresenta un'unica misura, gestita dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e presentata nel 2019 in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità, finalizzata a favorire e a sostenere idee, progetti ed iniziative capaci di attivare i giovani rispetto alle sfide sociali individuate come prioritarie per la comunità; a garantire l'uguaglianza di tutti i generi; a promuovere la creazione di nuove opportunità di partecipazione inclusiva alla vita economica, sociale e democratica per i giovani, anche al fine di favorire lo sviluppo e la crescita dei territori del Paese e soprattutto di quei territori caratterizzati da minori opportunità per i giovani, mediante l'agevolazione di progettualità a vocazione sociale. In relazione al terzo quesito, con il quale si chiede in cosa consistano i progetti di servizio civile da avviare al fine di garantire aiuto e assistenza alla comunità,

servizio civile universale, sono state disciplinate con apposite circolari tutte le iniziative necessarie per consentire al sistema di rispondere in maniera efficace alla crisi, continuando ad impegnare, nelle modalità ritenute opportune dagli operatori volontari della difesa non armata e non violenta della Patria, che costituisce la finalità principale del servizio civile. L'attività è stata svolta in costante raccordo con Regioni e Province autonome, con l'ANCI-Associazione nazionale Comuni italiani e con le rappresentanze degli enti di servizio civile e degli operatori volontari. In particolare, in coincidenza dell'inizio del *lockdown* sull'intero territorio nazionale, i progetti di servizio civile sono stati sospesi per circa un mese (dal 10 marzo al 15 aprile scorsi) e gli oltre 30.000 giovani operatori volontari sono stati considerati in permesso straordinario. In tale periodo, comunque, circa 3.400 volontari hanno proseguito il proprio servizio in quanto impiegati nell'ambito di organizzazioni che si occupano ordinariamente di soccorso e assistenza sociosanitaria, come Croce Rossa italiana, ANPAS, Misericordie d'Italia, solo per citare le principali, ma anche in molti Comuni. A partire poi dal 16 aprile, i progetti di servizio civile sono stati via via riavviati, dimostrandosi strumenti preziosi per garantire quotidiano supporto e assistenza alle comunità, in uno sforzo comune di solidarietà e di partecipazione in grado di incidere positivamente sul bene della collettività. Tale sforzo è stato reso possibile grazie al contributo dell'intero sistema di servizio civile e dal profondo senso dello Stato mostrato dagli enti e dagli operatori volontari, che hanno saputo reinterpretare il proprio impegno nel rispetto delle norme di precauzione che, seppur stringenti, rappresentavano un'imprescindibile necessità. La riattivazione progressiva dei progetti è stata attuata prevedendo accanto alla procedura ordinaria (ovvero secondo gli obiettivi progettuali originari) anche una procedura rimodulata (ovvero con obiettivi più o meno mutati e conseguenti nuove attività), attraverso modalità di svolgimento che potevano essere sul campo, da remoto o in maniera mista, combinando le due modalità. Al 16 aprile 2020, alla luce delle opportune valutazioni effettuate dagli enti e in accordo con gli operatori volontari, il 72 per cento dei progetti risultava riattivato con procedura ordinaria o rimodulata, a fronte del 28 per cento per i quali è stato necessario prevedere un'interruzione un'interruzione temporanea. Ciò significa che, già dal 16 aprile, 23.575 giovani (il 76 per cento del totale in servizio) sono stati riattivati. Soltanto 5.692 operatori volontari hanno dovuto fermarsi di fronte all'impossibilità di proseguire il proprio servizio nei progetti in cui erano impegnati, mancando le sufficienti condizioni di sicurezza o gli strumenti organizzativi ed operativi necessari a ripartire. Di questi 23.575 volontari, 13.044 (il 55 riprendevano le proprie attività sospese così come erano essenzialmente previste nei progetti originari, mentre 10.531 (il 45 per cento) risultavano impegnati in progetti che avevano subito una rimodulazione connessa alla situazione di emergenza. I prossimi progetti di servizio civile saranno avviati in via ordinaria all'inizio del 2021, in continuità con quelli attualmente in corso e con un inevitabile, leggero ritardo rispetto agli anni precedenti a causa dell'emergenza Covid-19. Il 29 maggio scorso è scaduto il termine per gli enti per la presentazione dei loro programmi di intervento che terranno dunque conto del nuovo contesto sociale ed economico che il Paese sta vivendo e si incentreranno prevalentemente su ambiti di azione connessi all'assistenza delle persone più fragili - compresi adolescenti e giovani che vivono in particolari situazioni di disagio ai processi educativi, agli scambi intergenerazionali, alla resilienza delle comunità. Tali programmi sono stati predisposti secondo quanto previsto dal Piano triennale 2020-2022 e dal Piano annuale 2020 per la programmazione degli interventi di servizio civile, piani che hanno il loro fondamento negli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, recepiti dalla nostra Strategia nazionale. In particolare, gli enti hanno presentato programmi tali da impiegare un numero di operatori volontari superiore ai 67.000; tali programmi sono attualmente in fase di valutazione da parte del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Le attuali risorse finanziare disponibili sul Fondo per il servizio civile universale, così come stabilito dalla legge finanziaria 2019, al netto dei tagli operati e con gli incrementi disposti dai decreti legge adottati con riferimento all'emergenza in atto, ammontano a circa 182 milioni di euro, cui si aggiungono 42 milioni di euro circa di residui dei precedenti esercizi, per un totale di circa 224 milioni di euro che potranno garantire poco meno di 41.000 posti, in linea con lo scorso anno. Grazie poi alle risorse provenienti dal Programma PON-IOG Garanzia giovani, pari a circa 53 milioni di euro, si potrà contare su 8.300 posti aggiuntivi che porteranno ad un contingente totale di circa di 49.000 posti. Ulteriori risorse consentirebbero di potenziare ancora questo importante istituto destinato ad attività preziose in un contesto delicato di post-fase acuta emergenziale, garantendo un più ampio finanziamento finanziamento dei programmi presentati per un numero maggiore di posti. Sarà necessario ricostruire il tessuto sociale del Paese, prestando particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili e in questo senso un investimento maggiore sul servizio civile si rivelerà un piano di azione di grande efficacia per i giovani. Sempre in relazione al terzo quesito, si segnala il progetto *Time to care*; un'iniziativa di *welfare* leggero rivolta ai giovani tra i diciotto e i trentacinque anni che rappresentano una risorsa fondamentale per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. Iniziativa finalizzata alla promozione di azioni di sistema sui territori in grado di favorire lo scambio intergenerazionale

il servizio civile è uno dei componenti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, organismo presieduto dal Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, che ha il compito di predisporre documenti ufficiali relativi all'infanzia e all'adolescenza, ulteriore sede di confronto e scambio di conoscenze, utile alla pianificazione di un piano generale per l'adolescenza.

Signor Presidente, apprezzo molto questa sua attenzione, che immagino sia legata anche all'importanza del tema. A tal proposito voglio ringraziare il Sottosegretario

nessuno può più far finta di non vederla, perché è come se lampeggiasse incessantemente. La crisi di questi mesi, che si sovrappone ad una crisi che infatti colpito più duramente chi è più indifeso, in particolare i giovani e le donne, e toglie fiducia e futuro alle nuove generazioni, che già più di tutti pagano politiche sbagliate e i guasti dei tagli al *welfare* al *welfare* municipale - al diritto allo studio e agli investimenti per il lavoro. Da troppo tempo si è inceppato il meccanismo che permette a chi viene dopo di avere più possibilità e da troppo tempo i figli hanno invece meno opportunità rispetto ai padri: questo è un tradimento dei fondamenti della nostra democrazia democrazia e del nostro patto repubblicano. Dobbiamo infatti rimuovere gli ostacoli che impediscono ad un giovane di andare avanti, ostacoli che questi mesi di *lockdown* hanno ingigantito, in una società con troppe porte chiuse, troppe difficoltà e respingimenti. Questi muri, in questi mesi, sono diventati ancora più insormontabili. È stato infatti un tempo di grande disorientamento per i più giovani in particolare per chi vive condizioni di marginalità e di esclusione. È come se si fosse rotto il meccanismo dell'adolescenza, che però è una fase esistenziale cruciale, che dobbiamo proteggere, è quella in cui molto spesso si decidono le sorti di un'esistenza. Adolescenti, bambine e bambini sono stati privati improvvisamente dei riferimenti del proprio mondo, innanzitutto della possibilità di andare a scuola, di stare con gli altri, di fare sport e socialità e questo per chi non ha famiglia ha significato perdere tutto, per chi vive una disabilità o un bisogno speciale è come se si fosse spenta una luce vitale. Nel pensiero di tanti nostri bambini e ragazzi improvvisamente è comparso il tema della sofferenza, della paura del contagio, della morte e dell'incertezza, entrato in modo prepotente, molto spesso causando un disagio psicologico. È come se questi mesi di blocco abbiano spezzato una dinamica di crescita individuale e collettiva, che è fondamentale non solo per le singole vite, ma per l'intera nostra società e per la sua capacità di progredire. Prima del Covid-19, 1.260.000 minori vivevano in condizioni di povertà assoluta, anche in conseguenza dello strascico della crisi economica del 2008. Oggi sappiamo che sono molti di più. Sono i più a rischio di dispersione, di abbandono scolastico e, quindi, di perdersi. Scuola chiusa ha significato anche mense e palestre chiuse e, quindi, il venir meno di pasti completi per molti, di una corretta attività motoria, di una mancanza di apprendimento, di salute e di nutrizione, che rappresentano un costo sociale altissimo e insopportabile. Questo ci dice che dobbiamo prendere coscienza di tutto questo come di una battaglia vitale per il nostro Paese e per tutti gli schieramenti. Per questo, chiediamo al Governo, con forza, un piano nazionale per l'adolescenza e per i giovani, che aiuti i più fragili a riprendere la strada, che prevenga e contrasti il disagio giovanile, che leghi inclusione e innovazione sociale, che dia più forza all'associazionismo giovanile, che rilanci il servizio civile universale come legame di comunità solidali, che sostenga lavoro e iniziative di imprenditorialità giovanile, che dia quella rappresentanza che alle nuove generazioni manca, quella voce che è troppo fragile nel nostro Paese. Signor Presidente, abbiamo il dovere di mettere le ragazze e i ragazzi del nostro Paese nella condizione di credere in se stessi, nel proprio talento, di essere protagonisti e di realizzare il progetto di vita e a questo fine avere anche i fondi necessari strategici, anche utilizzando

Presidente, onorevoli senatori, l'emergenza sanitaria derivante dal diffondersi dell'epidemia da Covid-19, che ha colpito duramente il nostro Paese, ha determinato, tra le altre cose, la sospensione di tutte le attività e le competizioni sportive. La linea del Governo è sempre stata, sin dal primo giorno, una linea prudenziale che ha messo al primo posto la salute di tutti i cittadini, anche e soprattutto di tutte le persone coinvolte nel mondo dello sport. Com'è noto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nel tener conto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, al fine di sostenere la graduale ripresa delle attività sportive, ha consentito, a partire dal 4 maggio 2020, le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Il Dipartimento per lo sport, già Ufficio per lo sport, ha emanato, in data 3 maggio 2020, le linee guida circa le modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali, documento redatto su impulso del CONI e del CIP, elaborato in stretta sinergia con la Federazione medico sportiva italiana, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, nonché validate dal Comitato tecnico scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione civile. Il suddetto documento ha previsto espressamente la previsione, in capo agli enti sportivi riconosciuti dal CONI o dal CIP, di emanare appositi protocolli di dettaglio, che tengano conto tanto delle indicazioni delle linee guida Generali, quanto delle specificità tecniche organizzative delle singole discipline. dei ministri del 17 maggio 2020 sono state consentite, altresì, le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti degli sport di squadra. Ciò ha rappresentato un primo passo verso la ripresa di tutti i campionati. Con procedimento analogo agli sport individuali, il Dipartimento dello sport ha prontamente emanato le linee guida generali, in data 18 maggio 2020. Prima che il Governo assumesse decisioni in ordine alla ripresa delle competizioni, va comunque ricordato che alcune importanti federazioni hanno decretato la conclusione anticipata definitiva della stagione 2019-2020. Si pensi, tra le altre, alla La ripresa dei campionati o la loro conclusione è dipesa dall'autonomia delle singole federazioni, a sostegno delle quali è stato introdotto, nel decreto rilancio, l'articolo 218, recante misure in materia di disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati professionistici

ha deliberato la volontà di riprendere e portare a termine i campionati professionistici delle serie A, B e C, sancendo, di contro, lo stop definitivo di tutti i campionati dilettantistici a partire dalla Serie D. A seguito dell'incontro tenutosi in modalità videoconferenza dall'autorità di Governo delegata in materia di sport con tutti i rappresentanti del mondo del calcio, in data 26 maggio è stata stabilita la ripresa dei campionati di serie A e B per il 20 giugno, previa definizione dei calendari da parte della Lega calcio, mentre la Lega Pro aveva prefigurato la possibilità di effettuare i *play-off* e i *play-out* salvo diversa posizione da parte del Consiglio federale. In data 28 maggio 2020 il comitato tecnico-scientifico ha dunque approvato il protocollo elaborato dalla FIGC e dalla Lega calcio calcio per la ripartenza delle competizioni. Si ritiene che il lavoro complesso e non privo di difficoltà che è stato svolto dal Governo con tutti gli altri soggetti coinvolti dal CTS FIGC abbia consentito di portare a termine il campionato di calcio della stagione 2019-2020 da poco concluso, destituendo di ogni fondamento le ipotesi richiamate in premessa dall'onorevole l'interrogante riguardo una presunta volontà di di non portare a termine i campionati di calcio. Siamo oggi impegnati affinché la ripresa della prossima stagione già alle porte possa avvenire in sicurezza e con graduale riapertura al pubblico qualora le condizioni generali dell'epidemia lo consentiranno. secondo quesito sull'indennità dei collaboratori sportivi per i mesi di aprile e maggio, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stata confermata l'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio (misure già previste nel decreto cura Italia per il mese di marzo) in favore dei lavoratori sportivi

Si tratta di un importante riconoscimento per una categoria spesso trascurata e poco tutelata che invece merita i giusti diritti e la doverosa attenzione. Con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 è stata ulteriormente prorogata l'indennità anche per il mese di giugno. Nonostante i provvedimenti adottati in merito alle misure di contenimento abbiano consentito la riapertura dei centri sportivi, la ripresa delle attività la ripresa delle attività sportive è stata molto graduale ed interi settori, quali ad esempio gli sport di contatto, non hanno potuto riprendere l'attività fino al 25 giugno 2020, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio

Sempre con il decreto cosiddetto rilancio, sono state introdotte ulteriori misure di sostegno, tra cui l'estensione del credito d'imposta previsto nel decreto cura Italia per i canoni di locazione dell'immobile ad uso non abitativo. La norma riconosce a vari soggetti, fra cui enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento in relazione al canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività istituzionali. Il beneficio è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio. In tema di canoni di locazione, com'è noto, l'articolo 116 e del decreto rilancio ha previsto la possibilità di rinegoziare i rapporti concessori tra enti locali e ASD-SSD che hanno in gestione impianti di proprietà pubblica al fine di ristabilire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, nonché la possibilità di rinegoziare i termini del contratto di locazione tra soggetti privati ai sensi del codice civile, prevedendo la corresponsione di un importo pari al 50 per cento della somma originaria pattuita. Infine, si ricorda altresì il credito di imposta per i lavori necessari ad adeguare gli immobili alle prescrizioni anti-Covid nella misura del 60 per cento, per un importo massimo di 80.000 euro per la sanificazione dei locali. terzo quesito sulle agevolazioni fiscali per ASD-SSD, il decreto cura Italia, ai sensi dell'articolo 61, comma 2, che ha modificato l'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, estendeva l'ambito di applicazione della sospensione fino al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavori dipendenti, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente alle federazioni sportive nazionali, agli

nonché ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli (lettera p). Con il decreto cosiddetto rilancio, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. L'articolo 97 del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 ha disposto, infine, il pagamento dei versamenti sospesi nella misura del 50 per cento al 16 settembre prossimo venturo, mentre ha ulteriormente prorogato il versamento del restante 50 per cento senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Inoltre, il suddetto provvedimento ha introdotto la misura del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo della sponsorizzazione

dei ministri del 17 maggio 2020, l'articolo 10 introduce uno specifico riferimento all'esecuzione e monitoraggio delle misure previste per il contenimento del contagio attraverso il coinvolgimento diretto delle prefetture. Le disposizioni di cui al suddetto decreto si applicano altresì alle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi Statuti e norme di attuazione. Premesso quanto sopra, mantenendo l'approccio prudenziale del Governo, è stato ritenuto quanto mai opportuno, al fine di favorire la ripresa delle attività e la ripartenza di tutti i settori, non solo quello sportivo, introdurre un *quid* decisionale alle Regioni relativamente agli sport di contatto. L'articolo 1, comma 1, lettera *g)* del

ha, infatti, previsto la possibilità di far ripartire gli sport di contatto dal 25 giugno ultimo scorso in quelle Regioni che, d'intesa con il Ministero della salute e l'autorità di Governo delegata in materia di sport, avessero accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento epidemiologico.

È stato nel contempo costituito un apposito comparto per operazioni di liquidità che consente l'ammissibilità a esso ai soggetti sportivi (Federazioni sportive nazionali ed Enti di promozione sportiva), che attualmente sono esclusi dall'accesso alle garanzie del Fondo centrale di garanzia per le PMI. Inoltre, è stato costituito un apposito comparto del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 1295 del 24 dicembre 1957, fino al 31 dicembre 2020, per le esigenze di liquidità dei suddetti organismi sportivi che saranno concessi secondo le modalità stabilite dal Comitato di gestione dei fondi speciali dell'istituto medesimo. Tali strumenti consentiranno di garantire 100 milioni di euro di finanziamenti a tasso zero e consentiranno, altresì, di ridurre tempi e oneri per chi ha necessità immediate di liquidità, al fine di poter far ripartire le attività e valorizzare l'importante ruolo sociale dello sport. Con l'articolo 217 del decreto rilancio, al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato istituito, nello nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale», le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo sport - già Ufficio per lo sport - per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. Il finanziamento del fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni per il 2021 ed è alimentato da una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere. In sede di conversione del suddetto decreto legge, il fondo è stato implementato di ulteriori 30 milioni di euro. Inoltre, è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa «Insieme per lo sport» tra Dipartimento per lo sport, la società Sport e Salute SpA, il CONI e il CIP i quali, ognuno in base alle rispettive disponibilità, hanno messo insieme risorse per circa 32 milioni di euro così ripartiti: 10 milioni Dipartimento per lo sport, 12 milioni Sport e Salute, 5 milioni CONI, 5 milioni CIP. Vale la pena in questa sede ricordare anche la pubblicazione, avvenuta il 20 luglio ultimo scorso, del bando di finanziamento pubblico «Sport e Periferie». Per l'anno 2020 sono stati stanziati 140 milioni di euro, che saranno destinati a interventi di ammodernamento e recupero dell'impiantistica sportiva in tutta Italia. La novità è che potranno accedere al fondo non solo gli enti locali proprietari degli immobili, bensì anche associazioni e società sportive che hanno impianti in gestione o di proprietà. Come descritto in risposta al primo quesito, le linee guida generali per la ripresa degli allenamenti individuali, in un primo momento, e degli allenamenti degli sport di squadra e dello sport di base, successivamente, predisposte dal Dipartimento per lo sport (già Ufficio per lo sport) hanno posto le basi per l'elaborazione degli specifici protocolli redatti dalle diverse federazioni che, una volta approvate dal Comitato tecnico-scientifico, hanno consentito la ripresa e la conclusione conclusione dei campionati.

al coinvolgimento delle generazioni e del pubblico negli eventi sportivi, che è un valore in sé e che, a mio avviso, dobbiamo assolutamente proteggere e garantire. Il tema centrale dell'interrogazione è rappresentato dall'incentivo che si vuole dare alla ripresa degli eventi sportivi con la presenza del pubblico. Questa è la sfida che ci poniamo nelle prossime settimane, tenendo conto del fatto che va assolutamente apprezzata la linea prudenziale adottata dal Governo sia nella fase di criticità massima dell'emergenza epidemiologica, quando è stato inevitabile sospendere le manifestazioni, quando c'è stato il coraggio di riprenderle, anche in una logica europea di ripresa dei campionati e delle attività sportive all'aperto più in generale. È quella la strada che dobbiamo perseguire. Sicuramente noi, come Governo, avremo linee guida contenenti i principi sulla base dei quali rilanciare gli eventi sportivi. Dovremo verificare, anche a livello europeo, come ripartirà tutto il sistema dello sport all'aperto, a partire dal calcio e non solo. Infatti, c'è tutto un insieme di sport non praticati all'aperto che coinvolgono

hanno consentito nei mesi di aprile, maggio e giugno di avere un *bonus* e un sostegno al reddito. Credo sia stato importante introdurre la norma che permette alle società sportive di ricontrattare i contratti di locazione e di e di concessione degli impianti, perché è chiaro che le condizioni economiche che potevano esserci, in termini di tesserati e magari, in qualche caso, anche di presenza del pubblico, prima dell'emergenza sono completamente cambiate. Quindi, sono giusti questo sostegno e questa attenzione. Credo ci sia quindi uno sforzo importante. Ciò che dobbiamo porci come sfida è consentire agli eventi sportivi di tornare ad avere il pubblico, che è l'aspetto che

Signor Presidente, passo a illustrare l'atto sulla cumulabilità delle indennità Covid-19 con i trattamenti pensionistici diretti. Preliminarmente è opportuno evidenziare che, come noto, la formulazione originale del cosiddetto decreto cura Italia non prevedeva la cumulabilità delle indennità Covid-19 con i trattamenti pensionistici diretti, incluso l'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge n. 222 del 1984. Su questo quadro normativo successivamente siamo intervenuti con il decreto rilancio. Quindi è oramai acclarato che l'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato e integrato dall'articolo 75 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al comma 1-*bis* ha espressamente previsto che le indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. con l'assegno ordinario di invalidità. nell'ambito della quale sono state fornite istruzioni operative. In particolare, l'istituto previdenziale ha preso in considerazione sia il caso di coloro che si sono visti rigettare la domanda per l'ottenimento dell'indennità Covid-19 esclusivamente in ragione della titolarità dell'assegno ordinario di invalidità, sia l'ipotesi dei lavoratori che non hanno affatto presentato domanda in quanto titolari del medesimo beneficio, prescrivendo rispettivamente che nel primo caso l'ente previdenziale avrebbe rivalutato *ex officio* le istanze originariamente presentate, accogliendole, mentre nel secondo caso ha indicato il termine finale entro il quale i richiedenti avrebbero dovuto presentare l'apposita istanza. Inoltre, nell'ambito dello stesso decreto-legge n. 34, in virtù dell'articolo 86, anche le indennità istituite ai sensi degli articoli 84, 85, 78 e 98, nonché il reddito di emergenza istituito dall'articolo 82 del medesimo decreto-legge, sono state ritenute cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. Da ultimo, voglio sottolineare che questa impostazione appare confermata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale stabilisce al comma 6 che le indennità a favore delle categorie previste ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo 9, ovvero lavoratori stagionali o dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dello spettacolo e altre categorie come i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA titolari di contratti autonomi occasionali incaricati alle vendite a domicilio (questo la dice lunga della frammentarietà del nostro mercato del lavoro), sono anch'esse cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Per quanto concerne la lamentata esiguità del trattamento pensionistico in questione e la richiesta di adeguamento dei relativi valori, evidenzio che il medesimo decreto-legge n. 104, all'articolo 15, è per dare attuazione a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 152 del 23 giugno 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38 della legge finanziaria 2002, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi ivi previsti (fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese, tredici mensilità, successivamente rivalutato fino a 651,51 euro per il 2020) sono concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, anziché ai soggetti di età superiore a diciotto anni. In particolare, la Corte ha affermato che il cosiddetto "incremento al milione", pari a 516,46 euro e successivamente rivalutato a 651,51 euro, da tempo riconosciuto per vari trattamenti pensionistici all'articolo 38 della legge n. 448 del 2011, debba essere assicurato agli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12

del sessantesimo anno di età attualmente previsto dalla legge. La medesima Corte ha stabilito che resta ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l'effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione. Di conseguenza, la maggiorazione sociale in questione è stata riconosciuta con effetto dal 20 luglio 2020 (data di pubblicazione) anche ai soggetti di età superiore a diciotto anni e fino ai cinquantanove anni che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità, di cui all'articolo 2 della legge n. 222 Concludo sottolineando la rilevanza della questione segnalata dalla senatrice Binetti, quindi posso assicurare che il Ministero che rappresento continuerà a mantenere alta l'attenzione sul tema affinché siano sempre garantiti i diritti e le condizioni spettanti a questi lavoratori.

a fronte - non se ne voglia - delle pensioni o comunque dei contributi che sono stati elargiti, a mio avviso in maniera in parte eccessiva e in parte ovviamente insufficiente, quando pensiamo per esempio al reddito di cittadinanza. Noi abbiamo davanti un invalido totale con una pensione di 286

Quindi nell'invalidità totale la condizione di disagio legata alla pandemia diventava ancora di più un ulteriore elemento di mortificazione, fino al punto di ridurre

compresa per esempio un'associazione molto particolare. Alle volte, infatti, quando si parla degli invalidi totali si pensa facilmente al cieco totale, cioè all'invalidità sensoriale e fisica magari dalla nascita, con tutta la gravità che questo presuppone,

non a una volontà di nuocere, ma al non aver studiato con chiarezza il problema a monte e al non aver evidenziato

hanno contribuito in qualche modo a ridurre questa ingiustizia. Mi auguro con tutto il cuore che se ne prenda atto per rivedere davvero tutto il pacchetto delle misure attraverso con cui ci si fa carico degli invalidi. Richiamo il rilievo che giustamente faceva presente il Sottosegretario

qualità della vita? Per di più abbiamo misure di stampo meramente assistenziale che non corrispondono né al bisogno né alla fattualità che viene posta in essere. Mi dichiaro

hanno tratto energie proprio dall'alleanza con le associazioni, o potremmo dire con una società civile che si sentiva penalizzata in questo senso; sul punto bisogna dare atto che un minimo di ascolto concreto lo hanno ottenuto.

Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti poiché con il loro quesito mi consentono di fornire chiarimenti in ordine a una questione interpretativa particolarmente complessa, in relazione alla quale mi scuso fin da ora se il linguaggio utilizzato non potrà escludere tecnicismi di natura giuridica. La questione oggetto dell'interrogazione attiene, infatti, al regime delle aspettative dei docenti e dei ricercatori nell'ipotesi di svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici e privati, o anche di direzione di enti, di istituti e di laboratori. In particolare, viene posto uno specifico quesito in relazione alla disciplina applicabile allo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici e privati, compresa la direzione di enti, istituti e laboratori. L'interrogazione, in sintesi, verte sulla presunta violazione dell'articolo 7 della legge n. 240 del 2010, nella parte in cui stabilisce una durata massima all'aspettativa in parola. In primo luogo, occorre subito chiarire che la norma, nel fissare un limite temporale di cinque anni, deve ritenersi applicabile alle sole ipotesi di aspettativa facoltativa, ovvero a quelle ipotesi per le quali la legge non prevede alcuna incompatibilità fra l'attività del docente o del ricercatore e lo svolgimento di altre attività. Di converso, l'aspettativa obbligatoria prevista dalla legge per le attività incompatibili con quelle dei docenti e ricercatori universitari, non può che non essere soggetta a limite temporale, poiché, come più volte affermato dalla Corte costituzionale, essa costituisce un istituto giuridico volto a garantire, in ossequio ai principi di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione, la partecipazione dei cittadini allo svolgimento di cariche pubbliche, in condizione di uguaglianza, riconoscendo ad essi la disponibilità del tempo necessario all'adempimento dei compiti propri degli uffici delle cariche pubbliche e, al contempo, la conservazione del posto di lavoro. Venendo al merito della questione oggetto dell'interrogazione, va innanzitutto precisato che, ai docenti e ai ricercatori che intendono assumere la presidenza o la direzione di enti, di istituti, di dipartimenti o di laboratori di ricerca, si applica, nel caso del CNR, in luogo del citato articolo 7, un regime giuridico di carattere speciale, previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 127 del 2003, non a caso rubricato «Disposizioni specifiche». Tale regime prevede che il professore o il ricercatore universitario, incaricati della presidenza del CNR, possano essere collocati in aspettativa obbligatoria, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Ne discende che per tali soggetti, in ragione della natura obbligatoria dell'aspettativa, non è ragionevole che si applichi il limite temporale previsto dall'articolo 7 della legge Gelmini, che, come detto, riguarda solo le ipotesi di aspettativa facoltativa. Invece, per quanto riguarda gli incarichi di direttore generale, di direttore di dipartimento o di direttore di istituto, la norma speciale di cui si è detto rinvia alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto del che non stabilisce alcun limite temporale. Ne discende quindi che, in virtù del carattere speciale di tale normativa, essa debba ritenersi prevalente rispetto alla disciplina generale prevista dall'articolo 7 della legge n. 240 Per tale ragione, il limite dei cinque anni stabilito dalla norma in questione può non ritenersi applicabile alle ipotesi evocate dagli interroganti. Inoltre, rispetto alla preoccupazione espressa dagli interroganti in ordine al presunto aggravio di oneri a carico della finanza pubblica, si rileva che le norme che disciplinano il regime di aspettativa obbligatoria e facoltativa prevedono che tali oneri, compresi il trattamento previdenziale e assistenziale, sono a carico degli enti pubblici che conferiscono gli incarichi di presidenza o di direzione ai docenti e ai ricercatori universitari collocati in aspettativa, circostanza, questa, che garantisce circa la neutralità finanziaria di tale istituto. Tanto premesso, per quanto le motivazioni suesposte debbano ritenersi ragionevoli e compatibili con il quadro complessivo delle disposizioni inerenti lo stato giuridico dei professori universitari, nonché rispondenti al più generale interesse pubblico all'individuazione delle migliori competenze per l'assunzione di incarichi di tale prestigio, il Ministero intende effettuare ulteriori approfondimenti di natura giuridica in ordine al miglior contemperamento dei principi di cui si è dato finora conto. Ciò posto, desidero rassicurare gli onorevoli interroganti che non si mancherà di dare informazione in relazione agli esiti di tale approfondimento, dai quali potranno originare, laddove ritenuto necessario, anche futuri interventi normativi.

perché l'incertezza che regna sulla materia oggetto di questo atto di sindacato ispettivo e su altri aspetti del mondo delle docenze universitarie non può, a mio avviso, continuare a passare sotto silenzio. Ritengo che il ministro Manfredi, sia perché non oberato dal carico che gravava sui predecessori, sia perché come ex rettore conosce perfettamente anche le anomalie del sistema, è la persona giusta per rimediare, sempre che lo voglia. Dico sempre che lo voglia perché, al netto della promessa di approfondimenti, che ovviamente apprezzo moltissimo,

come se quella fosse una *lex specialis* relativa al Consiglio nazionale delle ricerche, mentre è una norma generale dell'ordinamento universitario, significa voler ignorare che tale è - intendo norma generale - la legge n. 240 del

legge n. 240 del 2010 (rubricato «Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori») pone invece, come da lei ricordato, un limite massimo pari a cinque anni anche consecutivi, senza prevedere deroghe,

e organismi pubblici o privati (e tale è anche il CNR, come gli altri enti pubblici di ricerca). Il dettato normativo è abbastanza chiaro, eppure la non corretta applicazione dell'articolo 7 è costante, tanto è vero che per restare al CNR - ed era la ragione per la quale presentai l'interrogazione - dal luglio 2019 il consiglio d'amministrazione ha più volte assegnato scientemente incarichi di direttore di istituto o di dipartimento a docenti universitari che a quella data avevano già superato i quattro anni di aspettativa. Faccio qualche esempio: il professor Antonio Occhiuzzi, il professor Claudio Conti, il professor Salvatore Capasso, la professoressa Roberta Ramponi o il professor Giuseppe Gigli. Una situazione oggettivamente scabrosa, stante questa incertezza di applicazione della norma. Mi permetta però di fare anche un cenno ad altre criticità riguardanti la mobilità e le attività extrauniversitarie dei professori, di cui troppo spesso si tace pur avendole sotto gli occhi. Faccio due esempi, signor Presidente. È di questi giorni la condanna in primo grado per danno erariale dell'ex assessore della giunta regionale campana, ingegner Ennio Cascetta, per diverse consulenze svolte mentre era docente a tempo pieno all'Università Federico II. II. L'aver stralciato *in extremis* la settimana scorsa l'emendamento 19.15 al decreto-legge semplificazioni, presentato dai colleghi della Lega, ha dunque evitato che quei comportamenti diventassero improvvisamente leciti ed ha scongiurato una liberalizzazione totale che avrebbe reso molti docenti universitari del tutto sconosciuti agli studenti che frequentano i loro corsi, sublimando la mala pratica dell'affidamento esclusivo dell'attività didattica agli assistenti, a fronte di almeno duecentocinquanta ore che ciascun docente ordinario deve garantire al suo Ateneo. A questo proposito - passo a un secondo esempio, cambiando leggermente ambito - il professor Massimo Sanna, ordinario di archeologia classica all'Università Federico II ha preso quella docenza nel dicembre 2015, poco prima di lasciare la soprintendenza archeologica di Pompei, Ercolano e Stabia per assumere dal 4 gennaio 2016 il mandato di direttore di prima fascia responsabile del Parco e museo di Pompei, conferitogli anch'esso grazie a un comma 6, dunque a scapito della dirigenza interna del Mibact; un incarico a tempo pieno con contratto di diritto privato che comporta esclusività. Ebbene, il professore ha mantenuto la docenza sia nel primo sia nel secondo triennio della direzione museale di Pompei, salvo che del secondo ha svolto circa un anno, essendo stato appena nominato direttore generale dei musei dello stesso Dicastero, altro incarico a tempo pieno e fuori sede, oltre ad avere al momento l'*interim* di Pompei (non saprei dire bene a quale titolo). Il professore risulta in forza all'università Federico II anche per il 2020-2021. Dunque, per chiarezza, signor Sottosegretario, le chiedo la cortesia di approfondire a mo' di esempio il caso del professor Sanna. La sua è una messa in aspettativa d'ufficio, oppure facoltativa, oppure una supplenza a titolo gratuito o cos'altro? Sul portale dell'Università Federico II non sono riuscita a trovare alcuna informazione dirimente al riguardo. Glielo chiedo nell'interesse degli studenti, innanzitutto, ma anche degli altri docenti a tempo pieno dell'Ateneo napoletano e delle tante università dove si verifica... Credo, infatti, che occorra fare chiarezza su situazioni che, ripetendosi, alterano la percezione della normalità, rendendo altresì ben chiaro che i baronati universitari sono tutt'altro che scomparsi e troppo spesso possono contare sulla sussiegosa accondiscendenza di vertici ministeriali.

i quali indubbiamente hanno sofferto più degli altri loro colleghi le limitazioni imposte a tutta la popolazione nell'ambito dell'emergenza Covid-19. Va detto che la questione in oggetto ha rappresentato da subito una priorità del Governo dal momento che è risultata immediatamente chiara la necessità di individuare misure specifiche e tempestive per far fronte alle esigenze degli studenti universitari fuori sede e, più in generale, delle loro famiglie. Proprio in quest'ottica, il Governo ha deciso di intervenire in maniera importante nel cosiddetto decreto-legge rilancio. In conversione a tale decreto, infatti, grazie anche alla meritoria sollecitazione delle forze parlamentari, il Governo ha incrementato il fondo per il sostegno alle locazioni di ulteriori 20 milioni di euro, da destinarsi esclusivamente alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede. Tale misura invero viene ad inserirsi nel più ampio contesto di aiuti adottati in corso d'anno dal Ministero dell'università e della ricerca, che fin da subito ha assegnato un ruolo centrale alla tutela del diritto allo studio, nella piena consapevolezza che l'emergenza che stiamo vivendo purtroppo è in grado di originare o accrescere diseguaglianze che naturalmente non possono essere tollerate. In quest'ottica, allora, desidero ricordare che, nell'ambito dei fondi previsti per l'emergenza Covid-19, ulteriori 20 milioni di euro sono stati destinati agli studenti che necessitino di un contributo economico per l'acquisto dei dispositivi digitali e per i servizi per la didattica; 165 milioni di euro sono destinati all'esonero totale e parziale dalle tasse universitarie, estendendo in questo modo la cosiddetta *no tax area*; per le medesime finalità, inoltre, altri 8 milioni di euro sono stati riservati agli studenti dalle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Sempre al fine di promuovere il diritto allo studio universitario, infine, il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, è stato incrementato di 40 milioni di euro. A queste rilevanti misure di ordine economico, il Governo ha aggiunto, d'intesa con le Regioni, alle quali, devo rammentare, compete primariamente la materia del diritto allo studio, una specifica disposizione nell'ambito del cosiddetto decreto agosto, che va fortemente nella direzione della tutela degli studenti fuori sede. Mi riferisco all'articolo 33, comma 2, con cui si è introdotta una deroga a beneficio degli studenti universitari fuori sede che, a causa della situazione conseguente alla crisi epidemiologica, potrebbero vedersi pregiudicato lo *status* di studente fuori sede e, conseguentemente, la fruizione delle relative borse di studio. Con tale disposizione si prevede, infatti, sia per l'anno accademico in corso di conclusione, sia per quello che sta per iniziare, che il riconoscimento della condizione di fuori sede possa essere soddisfatta anche da chi prende alloggio nel luogo della sede del corso per un periodo inferiore a dieci mesi, condizione che ad oggi risulta indispensabile, ai sensi dell'articolo 4 del 9 aprile 2001, per l'ottenimento della borsa di studio e che, proprio in ragione della possibilità che essa sia venuta meno per via delle intervenute limitazioni alla libertà di circolazione, potrà essere soddisfatta anche da chi abbia alloggiato fuori sede per soli quattro mesi. Tale previsione normativa è stata dunque motivata dalla necessità di evitare che la grave situazione di emergenza vissuta dal Paese potesse in qualche modo pregiudicare una forma di aiuto agli studenti e alle famiglie, in molti casi ritenuta invece indispensabile. Concludo rassicurando l'onorevole interrogante sulla intenzione del Governo di voler proseguire nell'adozione di ulteriori iniziative volte a supportare gli studenti fuori sede,

per cui lo studente potrà frequentare il corso di laurea a seconda della propria posizione in graduatoria. Si troverà, quindi, ad essere studente fuori sede, pur vivendo in una città in cui c'è una facoltà di medicina, se in quella facoltà di medicina non c'è un posto disponibile e quindi dovrà optare

Penso a città come quelle in cui la sede universitaria diventa il punto di riferimento della vita cittadina; città in cui il numero delle persone che ci vivono cambia radicalmente nei periodi in cui ci sono le lezioni, gli esami, la frequenza degli studenti rispetto a quando non ci sono. Questo significa che il tema dello studente fuori sede investe molto una grande rete di proprietari di alloggi, che vivono e subordinano la qualità della loro vita alla possibilità che il bene alloggio affittato diventi per loro una fonte di mantenimento.

Tutto il tema dell'alloggio dello studente fuori sede meriterebbe una riflessione seria e una sorta di Commissione d'inchiesta per monitorare come si svolge la vita degli studenti.

Anche questo è un problema: molti di questi collegi sono stati in gravi difficoltà nell'ultimo periodo, perché la difficoltà della famiglia dello studente nel far fronte ai costi si è tradotta poi in una difficoltà sia delle famiglia locatarie, sia dei collegi e delle residenze in cui questi ragazzi si trovavano. È un tema composito composito quello che riguarda l'alloggio degli studenti. Giustamente, come diceva prima il sottosegretario De Cristofaro a proposito degli investimenti in strumenti di tipo digitale, è fondamentale

le loro famiglie e poi quella rete di servizi che si struttura intorno a loro e che è formata da una parte di famiglie locatarie, d'altra parte di collegi di merito o anche semplicemente di pensionati dove gli studenti possono raccogliersi. Garantire oggi le migliori condizioni possibili perché lo studente universitario sia concentrato a raggiungere il livello di eccellenza nello studio significa garantire non soltanto l'opportunità di portare a casa risultati significativi e positivi in termini di voto e quindi anche di accesso a potenziali potenziali borse di studio, ma anche di sviluppare quegli ambiti che li rendano idonei a intraprendere un'attività di ricerca o a partecipare a un dottorato di ricerca. Se lo studente non è concentrato sulla qualità del lavoro che sta svolgendo e non ha la consapevolezza forte di quel lavoro, lavoro, è una risorsa che perdiamo per il Paese intero. Ultima cosa e concludo: sappiamo che l'università non è solo un luogo di apprendimento, ma è anche un luogo di socializzazione, di relazioni e rapporti. Quindi, anche da questo punto di vista, facilitare queste strutture è veramente importante. Ringrazio e mi auguro davvero che tutto questo insieme di misure che appaiono molteplici, ma anche in parte anche frammentate (addirittura c'è il dubbio che lo studente conosca tutta la tavolozza delle opportunità che gli si presentano), abbiano un'organicità tale per cui sia facile sapere a cosa possono accedere e come, nei tempi più brevi e nel modo più efficace possibili. *(Applausi)*.

Signor Presidente, l'Italia segue con estrema attenzione l'*embargo* ONU sulle armi convenzionali all'Iran previsto dalla risoluzione 2231 del 2015 e in scadenza in ottobre. Lo fa in particolare la Farnesina grazie alle proprie rappresentanze diplomatiche all'estero e al coordinamento coi principali *partner* internazionali. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 15 agosto scorso ha bocciato la proposta di risoluzione presentata dagli Stati Uniti per il rinnovo dell'*embargo*. Stati Uniti e Repubblica Dominicana hanno votato a favore, mentre Russia e Cina si sono espressi in senso contrario e gli altri membri si sono astenuti. Pur non essendo membro del Consiglio di sicurezza, l'Italia condivide le preoccupazioni americane sulla scadenza dell'embargo. In linea con la posizione europea, riteniamo allo stesso tempo importante scongiurare una nuova *escalation* di tensione e la fine dell'Accordo sul nucleare iraniano. Nell'ambito dell'Unione europea, sulla base della decisione del Consiglio 413 del 2010, rimangono comunque in vigore, sino al 18 ottobre 2023, alcuni divieti di esportazione di determinate tecnologie di *software* e beni a doppio uso, l'embargo su armi e missili balistici e infine le sanzioni individuali per le persone fisiche e giuridiche designate, con le quali è di fatto preclusa ogni attività commerciale: tutte misure aggiornate e in linea con le determinazioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. A seguito della mancata approvazione della proposta di risoluzione sull'embargo di armi nel mese scorso, gli Stati Uniti hanno avviato la procedura per il ricorso al meccanismo di ripristino delle sanzioni onusiane preesistente all'Intesa sul nucleare iraniano, previsto dalla risoluzione 2231, istitutiva dell'Intesa stessa. La risoluzione prevede infatti che il meccanismo possa essere attivato dopo che uno Stato parte dell'Accordo sul nucleare abbia notificato un mancato adempimento significativo dello stesso Accordo da parte iraniana. Da ciò dovrebbe scaturire l'automatica riattivazione di tutte le sanzioni, a meno che non intervenga una risoluzione del Consiglio di sicurezza che decreti una nuova sospensione delle misure restrittive. Washington ha notificato il 21 agosto scorso alla Presidenza del Consiglio di sicurezza un non adempimento significativo dell'Intesa nucleare da parte dell'Iran. In seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU vi è tuttavia un parere pressoché unanime sull'assenza di legittimazione da parte americana a procedere, alla luce del ritiro di Washington dell'Accordo sul nucleare iraniano nel 2018. La Presidenza di turno mensile del Consiglio di sicurezza ricopre su questi aspetti un ruolo rilevante. Essa ha il compito di decidere se iscrivere o meno ai lavori dell'organo le richieste di attivazione del meccanismo. La Presidenza indonesiana di agosto ha ritenuto irricevibile la richiesta americana e l'attuale Presidenza del Niger non si è invece per il momento pronunciata. La posizione italiana al riguardo è in linea con quella espressa dall'Unione europea, sia direttamente dall'alto rappresentante Borrell che dal Servizio europeo per l'azione esterna, in qualità di Presidenza della Commissione congiunta dell'Accordo sul nucleare iraniano. Come annunciato nella Dichiarazione UE del 1° settembre, gli Stati Uniti non possono più invocare il meccanismo di ripristino delle sanzioni, essendosi ritirati dall'Accordo. In questa fase continuiamo a sostenere che la priorità vada attribuita a garantire la piena applicazione dell'Accordo sul nucleare iraniano: un pilastro dell'architettura di non proliferazione globale, in grado di contribuire alla stabilità regionale. Abbiamo quindi manifestato preoccupazioni per il progressivo disimpegno iraniano dall'Intesa sul nucleare e, sul fronte opposto, abbiamo salutato con favore la ripresa di una interlocuzione positiva tra Teheran e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, in materia di attuazione del Protocollo sulle salvaguardie. La missione in Iran del direttore generale Grossi, dello scorso agosto, è andata proprio in questo senso. Riteniamo fondamentale perseverare nella ricerca di un dialogo costruttivo con Teheran, un attore rilevante sul piano regionale, anche sui temi delicati come il futuro di lungo termine del nucleare, la proliferazione missilistica e il trasferimento di tecnologia balistica ad attori non statali.

risposta, ma mi sfugge qualche passaggio. Il Governo italiano concorda con l'alto rappresentante Borrell

È vero che restano in piedi delle altre sanzioni, ma è anche vero che le violazioni dell'Accordo sul nucleare, il JCPOA, sono sono state denunciate non dagli Stati Uniti, ma dalla stessa Agenzia nucleare delle Nazioni Unite. Dunque, servirebbe una posizione più chiara su questo aspetto,

esportatore di terrorismo. Si parla di 700 milioni di euro all'anno che vengono usati per finanziare il terrorismo internazionale. La stessa formazione di

svolga missioni di pace in parti del mondo e, dunque, era una formazione che andava in quella direzione. Rispetto al pericolo di un Iran nucleare, che viene perseguito, vantato e condotto in molti modi, da anni, dalle autorità iraniane, ci vorrebbe, da parte italiana (ed europea, certamente) un atteggiamento più chiaro e non così

un paio di altri Paesi hanno votato a favore del rinnovo dell'embargo e ha sottolineato che l'Italia non ha potuto votare perché, in quel momento, non faceva parte del Consiglio di sicurezza. All'inizio, mi era parso di capire che, se ne avesse fatto parte,

chieda il ripristino delle sanzioni riguardanti l'embargo di armi, alla luce delle violazioni dell'Accordo nucleare da parte dell'Iran. L'equidistanza non va bene. L'equidistanza fra chi esporta armi e terrorismo e chi cerca di contrastarlo non appartiene all'Italia. L'equidistanza tra il nostro principale alleato, gli Stati Uniti, e l'Iran, che da anni annuncia di voler distruggere uno Stato sovrano come Israele - che è nelle Nazioni Unite ed è riconosciuto dalle Nazioni Unite da prima dell'Italia - non è accettabile.

ringrazio il Sottosegretario per la risposta e per l'opportunità che dà a quest'Aula di sottolineare, ancora una volta, quanto il nostro Paese possa e debba avere un ruolo molto attivo rispetto alle enormi preoccupazioni che riguardano l'Iran:

sia dal punto di vista della funzione destabilizzante che svolge in tutta quell'area. Questo è esattamente il contrario della nostra impostazione di politica estera tradizionale, tra l'altro condivisa sempre, anche con cambi di maggioranza, dal Governo italiano. Per la nostra posizione nel Mediterraneo, per i nostri strumenti culturali, per le modalità con cui interveniamo da sempre nelle missioni internazionali, noi siamo, sul Medioriente, uno dei Paesi che svolge una funzione di stabilizzazione. Per questo sono soddisfatto, perché mi sembra chiara nella risposta la posizione del Governo italiano, che va nella direzione di rafforzare l'embargo, ma condivido quanto detto poco fa dal senatore Malan rispetto a due aspetti. Il primo è che possiamo e dobbiamo essere proattivi rispetto alle Nazioni Unite, rispetto ai Paesi membri del Consiglio di sicurezza e però membri anche dell'Unione europea; quindi, sempre di più devono riuscire a rappresentare l'intera Unione europea rispetto a quei seggi e farsi portatori di un embargo che - lo dico con grande chiarezza - non è la soluzione migliore al mondo. Non amo questo strumento e credo che dovremmo andare sempre di più verso sanzioni individuali sul modello del Magnitsky Act, approvato recentemente dal Governo tedesco, ci sono delle proposte di legge anche nel Parlamento italiano. Credo che dovremmo prendere in mano queste soluzioni, perché dobbiamo avanzare rispetto agli strumenti di condanna dei regimi che colpiscano sempre meno i popoli e sempre di più invece i colpevoli dei regimi, perché i popoli di quei Paesi rischiano di essere vittime due volte. Nel caso di un embargo rispetto alla vendita di armi, però, è evidente che non ci sono alcuna possibilità e alcuna valutazione secondo cui si possono vendere armi a un Paese che minaccia i Paesi confinanti e che interviene in maniera destabilizzante anche nella lotta al terrorismo, diventando uno strumento invece di promozione del terrorismo internazionale.

il Ministro della difesa e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Ministro, Giulia Schiff, giovane vincitrice del 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare, nel 2018 assume servizio presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli, supera l'esame di passaggio, volo da solista, e consegue quindi il grado di sergente pilota. Nella data del suo esame viene sottoposta al battesimo del volo, momento apparentemente giocoso, durante il quale viene però colpita con forti percosse; scossa e umiliata come donna e militare, invia le foto delle lesioni al padre, ex ufficiale dell'Aeronautica militare; il padre avvisa dell'accaduto un amico, ex collega di corso, alto ufficiale. In seguito Giulia riceve un drastico abbassamento della valutazione comportamentale, arrivando a subire sessantuno giorni di consegna. Successivamente viene proposta per l'espulsione dalla commissione di attitudine dell'Accademia. La Schiff sporge quindi denuncia alla procura militare nell'ottobre 2018. A seguito della pubblicazione in rete del filmato del rito, la vicenda assume rilevanza mediatica. Per questo, l'Amministrazione della difesa istituisce una commissione di inchiesta sommaria, le cui conclusioni non hanno riconosciuto responsabilità in capo ai quadri del comando. Il TAR del Lazio, nel marzo 2019, rigettava la domanda di reintegro, ma il Consiglio di Stato, con ordinanza successiva, reintegrava in via cautelare la Schiff come sergente aviere all'interno dell'Accademia per la prosecuzione del percorso percorso formativo. Nel frattempo le procure di Roma e Latina concludevano le indagini a carico di otto allievi del 124° corso per i fatti relativi al rito. Costoro, però, continuano a prestare servizio presso l'Aeronautica militare, senza che quest'ultima abbia mai preso alcun provvedimento a loro carico. Per il sommarsi di comportamenti discriminatori e punizioni disciplinari abnormi sia nel numero, che nel grado, la Schiff sporge denuncia - per *mobbing* questa volta - che si conclude però per insussistenza dei fatti. Sebbene reintegrata, il Comando scuole dell'Aeronautica militare negava alla Schiff la possibilità di pilotare e aggregarsi ai suoi paricorso. Il predetto divieto di volo è stato poi oggetto dell'ennesimo ricorso al TAR del Lazio, che, con ordinanza cautelare, ribadiva la legittimità dell'operato. Per i fatti di *mobbing* è stata presentata un'altra denuncia alla procura militare di Roma il 29 maggio scorso, con richiesta di inoltro alla procura ordinaria e a quella militare di Napoli, per quanto di competenza. Pertanto, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto; se, considerate le vicende descritte, non si possa rilevare una condotta discriminatoria e denigratoria ai danni di Giulia Schiff e, nel caso, se non ritenga necessario intervenire nei limiti delle attribuzioni,

di quanto accaduto potrà aversi solamente quando ne sarà conosciuto l'esito finale, voglio chiarire innanzitutto che qualsiasi comportamento lesivo della dignità personale non può essere tollerato. Passando al merito, ritengo utile mantenere distinti i diversi aspetti menzionati nell'atto di sindacato ispettivo. Mi riferisco a quello relativo al trattamento riservato all'allieva ufficiale pilota; a quello inerente al giudizio amministrativo da ella promosso, a seguito della sua dimissione dal corso per non attitudine militare, che - lo ricordo - è stata disposta in data 16 novembre 2018; e infine a quello riferito alla presunta condotta discriminatoria lamentata dall'allieva. Riguardo al primo aspetto, sono tutt'ora in corso gli accertamenti di competenza dell'autorità giudiziaria chiamata in causa - come correttamente evidenziato dagli interroganti - dalla stessa amministrazione militare in data 1° ottobre 2018, le cui conclusioni non potranno non essere tenute in debito conto nella susseguente valutazione disciplinare dei fatti. Riguardo invece al ricorso presentato dell'allieva il 23 febbraio 2019, a seguito della sua dimissione dal corso, il procedimento presso il TAR del Lazio è anch'esso pendente, con l'udienza per la trattazione del merito fissata per il prossimo 23 ottobre. Relativamente poi alla presunta condotta discriminatoria in particolare, all'asserito atteggiamento ostativo della Forza armata e infine alla possibilità di reintegrazione sostanziale dell'allieva, rappresento che l'Aeronautica militare ha ritenuto di dover procedere adempiendo alle determinazioni del giudice amministrativo.

assicurando il mantenimento del livello di preparazione acquisito nel corso precedentemente frequentato (cioè il 124°). Ciò nella considerazione che, come disposto dal Consiglio di Stato nella citata ordinanza - che cito testualmente - la prosecuzione e il completamento, con riserva, dell'attività formativa nel successivo corso (il 125°) risultano idonei ad assicurare l'interesse dell'allieva a non disperdere la maturazione dell'esperienza professionale e non determinano comparativamente profili di effettivo pregiudizio per l'interesse pubblico. Le disposizioni assunte quindi dalla Forza armata, allo stato, sono state giudicate congrue dall'ordinanza del TAR del Lazio n. 04377 del 18 giugno 2020, nelle more del giudizio sul ricorso tuttora pendente, nel merito, e che - come detto - si discuterà il 23 ottobre 2020 e delle cui delle cui determinazioni si terrà debito conto. In conclusione, onorevoli senatori, si tratta di una vicenda che seguo con doverosa attenzione, nella considerazione che non ci sarà comprensione per eventuali comportamenti che, anche alla luce dei pronunciamenti ancora attesi, si rivelassero difformi dagli imprescindibili principi di correttezza etica e professionale e di rispetto della dignità individuale.

pienamente convinta che così sarà - che i capi quadro, lei, signor Ministro, il Comando e l'Accademia militare, ciascuno con il proprio ruolo, prendano provvedimenti in tal senso, affinché tali pratiche vengano abbandonate e soprattutto cada quel velo di omertà che avvolge l'intero sistema militare e rende ordinario e normale ciò che non lo è. Così facendo, anche l'Esercito contribuirà in modo sostanziale a quel cambiamento culturale che sta avvenendo nella società civile e che si muove verso un nuovo modo di considerare il rispetto di genere, ma soprattutto della dignità della persona.

Signor Ministro, da una recente indagine giudiziaria bolognese condotta con grande professionalità - ma in corso evidentemente - è emerso uno spaccato preoccupante di diffusione di droga, cocaina in particolare, collegata allo spaccio e allo sfruttamento di minori. Questo è solo l'ultimo episodio di una catena di fatti analoghi che si stanno moltiplicando nel nostro Paese mentre - almeno a me - appare attenuata in maniera preoccupante l'attenzione della politica, del legislatore, delle autorità di Governo in ordine alla diffusione del fenomeno droga. Sembra un po' come se ci fosse un'assuefazione dell'opinione pubblica, una sorta di tolleranza silenziosa sul fatto che sostanze stupefacenti come le anfetamine, gli oppiacei, la *cannabis* e soprattutto la cocaina e loro derivati, nonché le nuove droghe sintetiche, siano ormai un elemento tollerato non solo tra le fasce di disagio sociale, ma anche e soprattutto fra i ceti più abbienti del nostro Paese. Spaccio, sfruttamento dei minori, traffico illegale naturalmente con connessioni nazionali e internazionali con la criminalità organizzata diventano tasselli di uno stesso mosaico, mentre praticamente non esistono più campagne di sensibilizzazione efficace e di prevenzione nelle scuole e nella società. Esiste per me anche un problema di innalzamento delle pene che può rendere più efficace il contrasto di questi fenomeni da parte delle Forze dell'ordine. Spesso, infatti, ci viene segnalato che coloro che sono coinvolti vengono immediatamente rilasciati e le conseguenze sono praticamente nulle.

l'onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere al fine della sensibilizzazione della società sulla problematica della diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani e se ritenga opportuno un intervento a livello normativo per contrastare il fenomeno. Va preliminarmente evidenziato che l'attenzione del Ministero dell'interno sul tema sul tema è da sempre elevata, nella piena consapevolezza che il consumo di tali sostanze può comportare gravi implicazioni per la salute e la vita sociale soprattutto dei giovani consumatori. Ritengo quindi che una strategia efficace per contrastare il fenomeno debba necessariamente includere politiche di prevenzione incentrate su attività d'informazione dei minori per diffondere una più alta consapevolezza dei pericoli per la salute e allo stesso tempo promuovere una più efficace sinergia tra Forze di polizia, mondo della scuola e famiglia. In questa direzione sono da tempo attive iniziative della Polizia di Stato per sensibilizzare il mondo scolastico attraverso campagne comunicative e informative finalizzate ad accrescere la consapevolezza dei giovani sui rischi derivanti dall'uso delle droghe. Nella stessa direzione è impegnato anche il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri con diverse progettualità che coinvolgono i *social media* e affidano anche alla realizzazione di un portale *web* la comunicazione sui rischi legati all'uso delle droghe in età scolare. Quanto all'attività di contrasto ai reati in materia di stupefacenti, soprattutto nella città di Bologna, informo che sia nel 2019 sia nell'anno in corso l'azione svolta dalle Forze di polizia ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e psicotrope e alla segnalazione all'autorità giudiziaria di diverse centinaia di persone con un incremento rispetto agli omologhi dati del 2018. In merito all'eventuale introduzione di nuove norme in materia, che naturalmente richiedono un'ampia concertazione con tutte le amministrazioni competenti, sono allo studio iniziative volte a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto, anche con riguardo ai casi di cosiddetta lieve entità, nonché a intervenire con efficacia nei confronti del crescente fenomeno dell'offerta di droghe sulle reti Internet, mutuando il meccanismo dell'oscuramento dei siti che diffondono materiale pedopornografico. ritengo soddisfatto della risposta del Ministro perché prima di tutto ha rassicurato - credo - il Senato e l'opinione pubblica sul fatto che non si sta con le mani in mano. Dicevo che il Ministero dell'interno è in un certo senso il semaforo: in questo caso credo che bisogna passare tra il giallo e il rosso; il verde è finito, ossia la tolleranza zero su questo fenomeno. tolleranza zero è fondamentale e il rapporto tra le Forze di polizia, la scuola e le famiglie, così come l'azione di contrasto in rete su Internet sono punti di una strategia per me ineludibile per il nostro Esecutivo. Devo dire che i dati che il Ministro ha riportato, seppure nella brevità di questa comunicazione - ovviamente sommariamente, e non poteva che essere così - ovvero il fatto che il Ministro abbia dichiarato che ingenti quantitativi sono stati individuati nel 2019 rispetto a quello che è successo l'anno precedente è già il segno che questo fenomeno non sta fermo, ma sta correndo. Lo spaccio

che le persone vengano arrestate al mattino e rilasciate la sera. Questo è assolutamente inaccettabile per l'opinione pubblica.

per far fuori la concorrenza. Oggi mi rivolgo a lei perché dai territori arrivano segnali preoccupanti su una ripresa delle attività classiche criminali. Oggi pongo l'attenzione sulla Provincia di Avellino. A San Martino Valle Caudina l'altro giorno c'è stato un omicidio le cui modalità sono quelle classiche di un delitto di camorra: i killer hanno ucciso con cinque colpi di pistola Orazio De Paola, cinquantotto anni, considerato dagli inquirente il principale referente del *clan* camorristico Pagnozzi, una delle potenti compagini criminali che controllerebbe tutti gli affari illeciti nella zona con robusti interessi anche nel basso Lazio, in Toscana e a Roma. In tempi *record* gli inquirenti hanno proceduto all'arresto con l'accusa di omicidio volontario del presunto *killer*. Ma quello che mi preme sottolineare qui è che negli ultimi tempi - come riportano gli organi di stampa c'è stata una pericolosa *escalation* con agguati e attentati ad Avellino: lo scorso 20 agosto davanti al parco Palatucci è stato ferito a colpi di pistola il pregiudicato Francesco Liotti, di trentaquattro anni, e dopo quarantott'ore è toccato all'abitazione, presa di mira con una "stesa", tipico raid armato camorrista; senza dimenticare gli attentati di Rione Mazzini e Valle, accadimenti che allarmano l'opinione pubblica e mettono a rischio l'incolumità dei cittadini. Lei sa bene, Ministro, che nella mia Regione, la Campania, sono state centinaia le vittime innocenti di camorra: sparano per strada e per strada spesso colpiscono gli innocenti. A intervenire oggi mi hanno spinto anche associazioni come Libera, impegnate per la legalità, preoccupate per questa *escalation*. Ecco, signor Ministro, perché siamo tutti preoccupati.

informo innanzitutto che le indagini della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ancora in corso, hanno consentito di acquisire già elementi di colpevolezza nei confronti di un pregiudicato arrestato nella giornata di ieri. In seguito a tale evento, sono state immediatamente intensificate le misure di vigilanza e osservazione, attraverso mirati servizi di prevenzione e controllo del territorio, anche tramite posti di blocco. Con riguardo, inoltre, al ferimento di un pluripregiudicato avvenuto sempre nel capoluogo irpino lo scorso 20 agosto, le indagini della competente autorità giudiziaria si stanno concentrando sull'accertamento della matrice delittuosa dell'episodio. Quanto al fenomeno di infiltrazioni camorristiche in Irpinia, ben rilevato anche nelle analisi criminali più recenti, assicuro che l'attenzione verso quel territorio è massima e che l'impegno delle Forze di polizia si traduce in un'intensa attività di prevenzione e di contrasto, soprattutto nella delicata fase che il Paese sta attraversando. allo specifico quesito rivolto dall'onorevole interrogante, informo che non si è mancato di valutare misure di potenziamento della rete di presidi della Polizia di Stato in Irpinia, che al momento possono contare su un numero complessivo di 455 unità. A breve sarà disposta l'assegnazione di un'ulteriore aliquota di 14 unità presso la questura e presso i reparti della Polizia stradale.

che parla proprio di una camorra moderna, silente e silenziosa, che ha i suoi rapporti con le amministrazioni pubbliche e infiltrazioni negli enti locali.

l'unico modo per evitare le partenze, gli sbarchi, i morti in mare, oltre che per azzerare il criminale commercio di uomini che registriamo purtroppo ogni giorno, ribadendo che in Italia si entra se si ha un permesso e se si ha un lavoro. Voglio brevemente ricordare che va anche fatta chiarezza sulle attività di certe sedicenti organizzazioni umanitarie ONG, che pretendono di svolgere la loro attività su navi straniere, che battono bandiera straniera, per poi scaricare solo sull'Italia il peso e il costo del loro intervento cosiddetto di soccorso per centinaia e migliaia di disperati. che esplicitamente, anche con arroganza, dichiarano di svolgere questa attività con finalità politiche, rivolte al contrasto delle forze politiche di destra sovraniste, che loro definiscono addirittura fasciste. L'alternativa a questa politica, cui anche lei ha fatto cenno, signor Ministro, è il caos che abbiamo visto e registrato in Sicilia negli *hotspot* e che ha determinato la reazione del presidente Musumeci. Ma c'è un'altra questione altrettanto grave, quella della rotta balcanica, che da almeno tre anni il sottoscritto, il mio partito e i consiglieri comunali da Tarvisio fino a Trieste stanno disperatamente cercando di porre all'attenzione del Governo e anche dei *media*. ogni notte da diversi anni attraversano clandestinamente quel confine decine e decine di persone sotto la regia di potenti ed efficientissime organizzazioni criminali. Queste persone non si sa che fine facciano e naturalmente ci sono problemi di ordine pubblico e sanitari che tutti possono intuire. Faccio brevemente riferimento ad almeno due problemi: uno è quello dei minori non accompagnati, che gravano per 100 euro al giorno su piccole amministrazioni comunali, che non sono in grado di sostenere questi pesi questi pesi economici enormi; l'altro è la situazione che si è determinata per esempio a Tricesimo, dove il sindaco del Partito Democratico ha dichiarato inaccettabile ed intollerabile la situazione per la quale immigrati in attesa anche del vaglio sanitario sono ammassati sul piazzale di un santuario avendo a disposizione un bagno chimico, una fontanella e passano le loro notti

le lamentele, le proteste e le preoccupazioni degli amministratori locali, delle autorità e anche della Regione. Le chiediamo in quanto tempo intenda intervenire e quali risposte intenda dare a queste grida di dolore.

e che stanno interessando parimenti il Friuli-Venezia Giulia per ciò che attiene alla rotta balcanica. Naturalmente si tratta di fenomeni ben distinti tra di loro, contrassegnati da cause diverse e con dimensioni certamente non comparabili. Riguardo alla pressione immigratoria su Lampedusa, gli sforzi italiani si sono concentrati nel ricercare la collaborazione delle autorità tunisine, in considerazione del fatto che il flusso più consistente proviene appunto dalla Tunisia in conseguenza della grave crisi politica e socioeconomica Grazie un'azione di contenimento efficace. È in ogni caso attivo, soprattutto con finalità dissuasiva, l'operazione Pelagie che vede impegnata l'Italia con assetti navali nel Mediterraneo centrale. Quanto alla situazione del Friuli-Venezia Giulia, il problema dell'incremento degli arrivi dalla rotta balcanica è stato affrontato anche con la collaborazione delle autorità slovene in virtù della quale è stato possibile incrementare il numero delle riammissioni e potenziare i servizi di controllo della fascia confinaria. Quanto al numero delle riammissioni, dal 1° gennaio al 7 settembre ultimo scorso sono da rilevare 874 riammissioni, Grazie a tale collaborazione si potranno vigilare meglio anche i valichi minori, che risultano più permeabili

di sindaci più esposti al fenomeno dei flussi e dei rintracci, specie dei minori non accompagnati, ha consentito di programmare una serie di interventi e misure tra i quali anche un incremento del già consistente contingente militare che opera in quella Regione nell'ambito dell'operazione Strade sicure (contingente aggiuntivo che arriverà nei prossimi giorni). intervenire in replica il senatore Ciriani, per due minuti. che queste interrogazioni, insieme a tutte le altre che ho depositato, servono a ricordare che noi non molleremo la presa su questo argomento così importante. Lei sa - e lo può chiedere agli uffici di polizia - che già nel 2018 c'era stata una triplicazione del numero dei fermati; nel 2019 un altro poderoso aumento delle persone bloccate al confine; nel 2020 - sono dati ufficiali, signor Ministro - solo nel mese di luglio e di agosto sono stati fermati al confine

confine va bloccato. Non serve distribuire i migranti, serve bloccarli al confine come fanno tutti gli altri Paesi sulla rotta balcanica, e servono accordi più stringenti con la Slovenia. Serve anche garantire spazi adeguati per confinare in quarantena queste persone, che non possono scappare dalla quarantena perché la gente ha paura e ha ragione ad averne, dato che alla caserma Cavarzerani di Udine, che ospitava seicento persone, ci sono stati tafferugli, incendi e fughe che la polizia ha dovuto reprimere. Quindi, signor Ministro, il tempo delle promesse è finito, la pazienza è finita. Lei credo possa rendersi conto, anche dall'incontro che ha avuto, che gli amministratori friulani e giuliani non sono persone abituate a gesti clamorosi, però ormai, come dicevo, la pazienza è finita, dunque se non arriveranno risposte chiare, forti e precise credo che gli amministratori potranno e dovranno utilizzare tutti gli strumenti giuridici e politici a loro disposizione per tutelare se stessi e per tutelare i diritti dei cittadini a vivere in sicurezza.

Invito i senatori a rispettare rigorosamente i tempi. [DAL Comunque, la sostanza è questa: i numeri parlano chiaramente. Signor Ministro, mi corregga se sbaglio, ma mi pare che i dati del suo Ministero dicano che quest'anno gli sbarchi - e parliamo di sbarchi - siano stati oltre 20.000, cifra che è pari esattamente a quattro volte quella dell'anno precedente, quindi siamo ritornati ai livelli del 2018. Non sono qui per fare propaganda agli amici della Lega perché si arrangiano da soli,

che stiamo un po' brancolando nel buio. Lei è venuta l'altro giorno a Trieste, come anche nel mese di luglio. Mi sembra che le risposte che il Governo continua a dare siano le stesse e siano balbettanti. siano balbettanti. È necessario ma non è sufficiente ciò che si sta facendo. Abbiamo bisogno di maggiore attenzione, abbiamo bisogno di maggiori tecnologie per controllare i nostri confini e qui il Governo deve decidere cosa vuole fare. Credo che dal punto di vista delle autorità regionali l'impegno sia massimo. È notizia di ieri che la prefettura di Udine ha messo a disposizione due pullman perché trenta immigrati provenienti dalla rotta balcanica risultavano positivi al Covid. Non sappiamo dove tenerli, non sappiamo che farne. Questo è il problema.

desidero preliminarmente evidenziare che il Ministero dell'interno ha una particolare attenzione al fenomeno dei flussi migratori verso il Friuli-Venezia Giulia, come testimonia anche la recente visita a Trieste in cui, proprio per trovare delle soluzioni concrete alle difficoltà organizzative e logistiche rappresentatemi *in loco*, ho incontrato il Presidente della Regione e un nutrito numero di sindaci. Quanto alla dimensione del fenomeno, preciso che l'intensa attività di polizia, rivolta al rintraccio di migranti irregolari nel territorio, ha consentito di attivare, molto più che rispetto al passato, le procedure speditive di riammissione verso la Slovenia. È una collaborazione questa con le autorità di oltreconfine che si basa sul rilancio dell'accordo del 1996 e che ha consentito di ottenere, come accennavo prima, risultati quadruplicati in termini di riammissione rispetto allo scorso anno. La collaborazione con la Slovenia potrà poi conseguire risultati ancora più efficaci sia tramite azioni congiunte di pattugliamento sia attraverso programmazioni coordinate dei servizi di controllo del territorio, specie nella vigilanza dei valichi minori. Inoltre, potrà sicuramente giovare, come dicevo prima, un incremento del contingente militare già operante in Regione, pari attualmente a 375 unità di personale dell'operazione Per quanto attiene alle misure di prevenzione del contagio da Covid-19, sono continue le interlocuzioni tra prefetti e amministratori locali allo scopo di garantire la sicurezza sanitaria dei cittadini. In esecuzione dei protocolli sanitari vigenti, tutti gli stranieri, al momento del loro ingresso nel territorio nazionale, sono sottoposti a tampone e alle conseguenti azioni di isolamento e quarantena a seconda degli esiti dell'accertamento. Per l'esecuzione di tali misure di prevenzione i prefetti delle province del Friuli hanno individuato diverse strutture che presentano le necessarie caratteristiche di sicurezza e sorvegliabilità.

che deve probabilmente il suo prestigioso incarico che ha svolto alla conoscenza che ha dei problemi e deve mediare tra due forze politiche che hanno due visioni diverse. Immagino che non sia facile. Nel 2016 si disse che la rotta balcanica era chiusa per un accordo che l'Europa fece con Erdogan; ciò fruttò alla Turchia circa 3 miliardi di euro.

Non è sufficiente dire che abbiamo aumentato ed intensificato i rapporti con la Slovenia perché li riportiamo in Slovenia. Cosa stanno facendo in Slovenia? Qual è la visione dell'Europa rispetto a questo dramma che è epocale, che ovviamente non riguarda solo

secondo Frontex, ci sono circa 100.000 persone, disperate, che stanno cercando di arrivare in Europa e passeranno attraverso il Friuli e la rotta balcanica; 8.000 sono già in Bosnia. Rispetto a questo, dopo quello che ci ha detto lei, non sono affatto tranquillo.

"sebbene ci sia una tendenza in aumento degli sbarchi autonomi rispetto al 2019, i numeri attuali non rappresentano un'emergenza. Le difficoltà sono di carattere logistico legate alle misure di profilassi sanitaria stabilite per il Covid

che ovviamente il Governo tiene nascosta, non differente rispetto a quelle che si possono trovare in alcuni centri del Nord-Est. Se ci fossero stati al Governo Matteo Salvini e la Lega, avreste chiamato i caschi blu ad intervenire: è una situazione che descrivere come indecorosa è dir poco.

a quanto ammonta il numero complessivo dei migranti approdati sulle coste di Lampedusa, dalla data di dichiarazione dell'emergenza sanitaria nazionale ad oggi, e se il Governo abbia intenzione di mettere in atto un piano che blocchi il continuo arrivo di imbarcazioni sulle nostre coste, ovvero se abbia in programma di continuare una politica di accoglienza indiscriminata l'aggettivo «indiscriminata», intendendo che oggi sono tunisini, che nulla c'entrano con i profughi o con chi viene dalle zone di guerra - nonostante l'aggravante dovuta alla gestione dell'emergenza sanitaria nel nostro Paese. se il Governo abbia intenzione di attuare un piano concreto in materia di contrasto all'immigrazione clandestina, che preveda anche un deciso intervento contro la tratta di esseri umani, che avete fatto riattivare. I numeri parlano chiaro! *(Applausi)*. sono quattro volte i 5.000 dell'anno precedente e sono esattamente, come già è stato anticipato, lo stesso numero del 2018. Quindi avete riattivato il meccanismo del traffico degli esseri umani. Chiedo come il Governo intenda gestire tutti i migranti attualmente ospitati sulle navi per le misure di isolamento dovute al Covid-19 una volta terminata la quarantena e se sia previsto un programma di rimpatrio per tutti coloro che non provengono da zone di conflitto o teatro di guerra. È evidente, signor Ministro, che l'*escamotage* che avete trovato in queste settimane di riempire con i migranti le navi traghetto, ovvero le navi da crociera, quando terminerà il periodo di quarantena cesserà. Sappiamo benissimo che dovete dare delle risposte e abbiamo già capito, come avete detto, che il vostro criterio è quello dell'accoglienza diffusa e ciò significa rimettere in moto quel meccanismo di *business* sulla migrazione, che noi abbiamo smontato. signor Ministro, la situazione che ho visto a Lampedusa e a cui facevo riferimento prima è anche quella di dieci carabinieri messi a controllare 360 sbarcati, che non avevano fatto il *test* per il Covid da più di una settimana. I carabinieri e i poliziotti non avevano neanche un posto in cui poter fare i propri bisogni

determinate da fattori geopolitici, che comportano la necessità di strategie articolate, nel presupposto che il confine italiano nel Mediterraneo rappresenta la frontiera esterna dell'Europa. Per questo motivo dobbiamo dare ancora più forza alle conclusioni del Vertice di Malta, del settembre dell'anno scorso, prevedendo un meccanismo strutturato di ripartizione obbligatoria applicabile a tutti gli Stati dell'Unione. Su questo siamo fortemente impegnati a costruire il necessario consenso a livello europeo e puntiamo a farlo nella cornice del nuovo Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo. Accanto alla strategia dei tavoli europei, intratteniamo relazioni bilaterali con Libia e Tunisia e le recenti missioni a Tunisi, che hanno visto il coinvolgimento dei commissari Várhelyi e Johansson, sono servite a rafforzare l'azione italiana ed europea di collaborazione verso quel Paese. Venendo alle specifiche domande, preciso che, dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza per l'epidemia, sono giunti a Lampedusa circa 12.000 migranti, la maggior parte dei quali tunisini, a riprova del fatto che un eccezionale elemento di spinta è costituito dalla crisi politica e socio-economica che ha investito quel Paese, anche per effetto della pandemia. Di fronte a una ripresa piuttosto intensa degli sbarchi, sono stati riattivati, al termine del *lockdown*, grazie alla collaborazione con le autorità tunisine, i rimpatri verso quel Paese, tramite due voli *charter*, per 40 migranti a volo. Informo, inoltre, che, anche a scopo dissuasivo, è stata attivata l'operazione Pelagie, che vede impegnati, con i rispettivi assetti navali, la Marina militare, la Guardia costiera e la Guardia di finanza, nella sorveglianza del tratto del Mediterraneo centrale interessato dai flussi. In merito, infine, alla gestione dei migranti al termine del previsto periodo di quarantena, la loro destinazione sarà conseguente al rigoroso accertamento del loro diritto a permanere nel territorio nazionale. Ministro dell'interno Matteo Salvini con la Lega al Governo: i flussi di immigrazione clandestina precipitano; torna al Governo il Partito Democratico e i flussi sono sostanzialmente quelli del 2018. Dopodiché, signor Ministro, le dico una cosa: vada a Lampedusa, ma ci vada non avvisando prima; ci vada durante una giornata qualsiasi di sbarchi. Ieri sera avrebbe trovato la gente esasperata ferma al porto, perché ieri sera stavano riempiendo ancora l'*hotspot* con gli ultimi arrivi. E quelli che voi chiamate «barchino», ovvero sbarchi fantasma, se lei va al porto, vedrà che sono barche con motori da 15 cavalli che non sono in grado di attraversare il Mediterraneo. Ma lei lo sa benissimo, perché i *dossier* dei Servizi li avete al Ministero: barche vengono da navi madre: sono portate a poche miglia dalla costa e poi sganciate. Lì va fermato il traffico degli esseri umani! *(Applausi)*. Se non intervenite su questa azione, vuol dire che voi avete scientemente deciso di rimettere in moto il traffico e il *business* degli immigrati clandestini, che, quando arrivano sul nostro territorio, costano agli italiani 600 milioni di euro. Su questi temi noi non siamo allora d'accordo e siamo molto preoccupati, signor Ministro, perché, anche dalle sue parole, si evince che il clima preelettorale sta facendo insabbiare tutte le informazioni. Volete smontare il decreto sicurezza, non sapete fermare gli sbarchi, non date risposte su dove ricollocherete chi si trova attualmente sulle navi quarantena. Quando sarà terminata la quarantena, che fine faranno quelli che hanno firmato semplicemente con una crocetta, sostenendo che sono richiedenti asilo? Gente che viene dalla Tunisia e che abbiamo visto, nei giorni scorsi arrivare con il cane al guinzaglio. Quelli li immetterete nuovamente nel meccanismo del *business* delle false cooperative in Italia? Queste cose noi ve le impediremo!

È una bella notizia, una notizia da noi di Italia Viva invocata da tempo. Siamo contenti che si proceda, ma è chiaro che, vista la situazione, bisogna essere consapevoli del rischio e della possibilità che, alla riapertura, si verifichino singoli casi di contagi, proprio a causa della contagiosità, ancora in atto, della pandemia coronavirus. Questo, però, non deve essere l'alibi per ulteriori slittamenti delle riaperture, ma deve essere, semmai, l'occasione per mettere in campo, innanzitutto, tutta una serie di misure stringenti, finalizzate al rinfocolarsi di nuovi contagi in secondo luogo, misure che consentano, appunto in via preventiva, di supportare anche le famiglie rispetto alla capacità di affrontare eventuali contagi dei propri figli e superare con tranquillità la situazione. infatti che, nelle indicazioni date dall'Istituto superiore di sanità, si prevede che, qualora si dovesse verificare il contagio anche solo di un alunno,

se intenda mettere in campo misure straordinarie, proprio in vista della riapertura delle scuole; se ci sia la corrispondente copertura finanziaria per le misure che intende predisporre; e, contemporaneamente, anche alla luce del pregresso, se non sia opportuno prevedere anche meccanismi idonei ad evitare casi di inopportuno abuso delle misure stesse. PRESIDENTE.

per fronteggiare l'emergenza sanitaria sin dal primo insorgere e la conseguente sospensione delle scuole e dei servizi per l'infanzia, il Governo ha messo in campo una serie di misure straordinarie a favore delle famiglie, quali ad esempio i congedi parentali straordinari e il *bonus baby sitting.* In considerazione del protrarsi dell'emergenza, il decreto rilancio ha ulteriormente rafforzato tali misure prorogando a trenta giorni il periodo di congedo ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione. Tuttavia, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, che è stata indicata come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione e nel settore privato, è stato altresì configurato come un vero e proprio diritto per i genitori lavoratori con i figli fino a Nell'imminenza della ripresa dell'anno scolastico, alla luce dell'andamento epidemiologico e delle indicazioni dell'Istituto superiore di sanità dello scorso 28 agosto, si è ritenuto opportuno intervenire nuovamente con norme *ad hoc* per gestire possibili necessarie assenze dei genitori lavoratori in caso di contagio o quarantena dei propri figli per effetto di contatti scolastici. scolastici. Per tale motivo, nel decreto-legge che è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* lo scorso 8 settembre, valido dal 9 settembre, si è introdotta una norma che prevede che, nel caso in cui il figlio minore fino a quattordici anni sia sottoposto alla misura della quarantena, il genitore per tutto questo periodo possa usufruire e far ricorso al lavoro agile, quando sia compatibile con le previsioni specifiche del lavoro pubblico e del lavoro privato. Ove tale prestazione lavorativa sia incompatibile con la modalità prevista agile, si potrà invece far ricorso - sempre per lo stesso periodo di quarantena - al congedo straordinario retribuito al 50 per cento e coperto da contribuzione figurativa. Per evitare ogni possibile abuso dei benefici, la norma dispone che le agevolazioni non possano essere utilizzate contemporaneamente da entrambi i genitori, ma questo anche nell'ottica di promuovere una maggiore corresponsabilità tra i padri e le madri. Per quanto riguarda la copertura della spesa, il beneficio dell'indennità è riconosciuto nell'ambito di un limite di 50 milioni di euro per il 2020, che risulterebbe tale da garantire la copertura di 50.000 casi con riferimento ai lavoratori dipendenti. In conclusione, voglio quindi assicurare la massima attenzione mia e di tutto il Governo per le problematiche dei genitori lavoratori e degli studenti e mi impegno sin d'ora, poiché la situazione epidemiologica è in continua evoluzione, ad avere cura attraverso i miei uffici di monitorare nuove esigenze delle famiglie che potrebbero nel caso insorgere e di intervenire qualora fosse necessario gli opportuni aggiustamenti.

sia importante da parte del Governo mettere in campo misure in via preventiva idonee a garantire la ripresa dell'anno scolastico nel modo più tranquillo possibile; quindi che, da un lato, si premurano di intervenire tempestivamente laddove si dovessero verificare casi di contagio e, dall'altro, mettano le famiglie nella condizione di poter programmare anche la propria attività

all'emergenza, ma anche di pensare ad un Paese più moderno, che veda anche un protagonismo femminile nel mondo del lavoro e che cerchi anche di favorire la conciliazione tra mondo del lavoro e mondo familiare in una gestione più equa tra uomo e donna.

14 agosto 2020, n. 104, istituisce e finanzia in ragione di tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 il Fondo per la formazione personale delle casalinghe. Il comma 2 del medesimo articolo rinvia a un successivo decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, la determinazione dei criteri e delle modalità di riparto.

rispetto alla media europea e sa anche che per affrontare e seriamente concretamente questo dato bisogna avere una politica di *empowerment* e di *mainstreaming*, cioè di capacità di politiche orizzontali. Non le sfugge che con questi dati si crea anche qualche problema rispetto al fatto che in questo decreto si parla di casalinghe. Voglio anche sottolineare un dato dal punto di vista proprio degli stereotipi. Le pare possibile che ancora nel 2020 parliamo di «casalinghe» quando anche i dati dell'Istat ci parlano di donne e di uomini? Non mi riferisco solo a donne che dopo il Covid, purtroppo, hanno avuto un incremento ulteriore di disoccupazione, ma anche al fatto che lavoriamo a una condivisione delle responsabilità familiari. È scoraggiante, per quei giovani mariti e padri che, invece, negli ultimi anni si sono affacciati alla responsabilità della condivisione anche dei lavori di cura. Credo che anche da questo punto di vista sarebbe importante

che lei dovrà adottare darà priorità all'utilizzo del fondo per la promozione di attività di formazione che siano funzionali all'inserimento lavorativo delle donne casalinghe e dei casalinghi, nonché all'obiettivo di valorizzare attraverso i servizi i lavori di cura, cioè costruendo davvero un'economia della cura. *(Applausi).*

qualificazioni e quindi strumenti di *empowerment* per rafforzare le proprie competenze. Lo scopo principale è evitare che la scelta di restare a casa diventi obbligata obbligata per la mancanza di alternative, garantendo alle donne quella libertà necessaria di scegliere e quindi di avere l'opportunità di accedere al mondo del lavoro. Si tratta, inoltre, anche di un'occasione per costituire reti di relazione che coinvolgano quelle donne che, a volte, vivono situazioni di isolamento e di solitudine che ne aggravano la situazione personale. Infine, c'è l'obiettivo, che è stato ricordato, di qualificare la condizione della cura nell'ambito di una maggiore condivisione tra la responsabilità maschile e quella femminile. Ricordiamo che certamente le donne oggi sono i soggetti su cui ricade maggiormente la cura domestica. Questa situazione si è ulteriormente aggravata a seguito della recente epidemia da Covid-19, per la quale le donne hanno pagato un prezzo altissimo, anche in termini di perdita di occupazione per il carico di lavoro e di cura non retribuito, che va a acuire una situazione strutturale che rischia di aggravare marginalità, fragilità e discriminazione. Per comprendere ancora meglio il peso del lavoro di cura sulla vita delle donne in particolare nel nostro Paese, è utile considerare un altro dato: la percentuale di donne inattive per responsabilità familiare sul totale della popolazione femminile e non solo su quella inattiva. L'Italia è il Paese dell'Unione europea con più donne inattive per responsabilità di cura. Riconoscere, quindi, un diritto alla formazione anche per le casalinghe e provvedere a investire risorse perché possano incrementare le loro competenze vuol dire garantire quei necessari diritti di *empowerment* garantiti

Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per portare a conoscenza dell'Assemblea un caso emblematico della situazione reale della scuola italiana a quattro giorni dall'apertura, prevista per il prossimo 14 settembre, al di là delle dichiarazioni del *premier* Conte e del ministro Azzolina.

di rinviare l'apertura dal 14 al 24 settembre, mettendo nero su bianco i motivi. In primo luogo, non ci sono i banchi

Questo fa particolarmente male perché il preside ha detto chiaramente che non se la sente di riaprire se non può garantire a tutti i suoi studenti - in particolare a quelli più fragili e portatori di *handicap*